vorrei annunciare, previa conferma da parte della Presidenza che tutti i Gruppi hanno ritirato gli emendamenti al decreto-legge

Quindi, ritira tutti gli emendamenti tranne uno? Sulla premessa la Presidenza non è in grado di pronunciarsi, allo stato.

intervenire in questa discussione per sottolineare di certo alcuni degli aspetti più positivi che contraddistinguono i i due decreti-legge che la Commissione bilancio ha esaminato ed emendato in 25 punti, e portato all'attenzione di questa Assemblea. Un lavoro di cui voglio ringraziare anzitutto il relatore, il senatore Silvio Lai, tutta la Commissione bilancio per l'impegno profuso, anche in tempi molto stretti, nell'esame di un provvedimento corposo, che risponde in modo concreto Grazie, dal susseguirsi di drammatici eventi, prima alla fine del mese di agosto e successivamente alla fine del mese Abbiamo visto quanto, all'indomani di quelle terribili scosse, il sistema nazionale di Protezione civile abbia saputo rispondere ancora una volta con efficienza ed efficacia già dai primi momenti successivi ai diversi sismi che si sono verificati, dimostrando di essere, agli occhi della comunità nazionale ma anche internazionale, internazionale, un fiore all'occhiello del nostro Paese. Credo che a tutto il sistema nazionale di Protezione civile debba andare il nostro più sentito ringraziamento. Mi è dispiaciuto ascoltare in quest'Assemblea parole a dir poco sconcertanti da parte di alcuni colleghi rispetto al giudizio espresso sulla capacità del sistema nazionale di protezione civile di corrispondere alle aspettative e ai bisogni dei cittadini colpiti dal sisma. Un sistema articolato, che fa capo al capodipartimento nazionale di protezione civile che coordina una serie di soggetti, ovviamente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma anche il sistema di volontariato e di protezione civile. PRESIDENTE. Colleghi, non è possibile lavorare con questo brusio. Vi pregherei di

dei vigili del fuoco, il sistema degli enti locali e delle colonne mobili di protezione civile che fanno capo alle Regioni, il sistema del volontariato nazionale di protezione civile, civile, che abbiamo visto in modo tempestivo giungere fin da subito nei Comuni colpiti dal sisma. Credo che per queste ragioni

il commissario governativo alla ricostruzione, Vasco Errani, che hanno proceduto congiuntamente, cercando, da un lato, di dare immediata assistenza alla popolazione e, dall'altro, legando le risposte all'emergenza e al percorso della ricostruzione. Ciò per consentire un pronto ritorno alla normalità per cittadini e imprese e per dare avvio alle prime fasi delle sistemazioni temporanee, a partire anche dalle verifiche sulle agibilità che determineranno la fase successiva della ricostruzione. crediamo il Governo abbia operato e stia operando bene e che oggi, attraverso l'approvazione di questo importante decreto-legge, serva mettere nelle mani del Commissario straordinario, dei cinque Presidenti di Regione e dei Sindaci in qualità di subcommissari, di subcommissari, strumenti maggiormente adeguati e corrispondenti alle aspettative, così come il decreto si prefigge di fare, oltre che le risorse

in campo, prendendo il meglio da quelle esperienze e innovando ulteriormente con l'idea che attraverso questo lavoro si possa migliorare anche la capacità con la quale le comunità locali messe nelle condizioni di rispondere alle aspettative dei propri cittadini e delle proprie imprese. Vi sono, a mio avviso, cinque imperativi a cui questo decreto si è ispirato. Il primo Il primo è la qualità massima dell'efficienza degli interventi, con il massimo rispetto possibile dell'identità dei luoghi e degli edifici.

Il secondo imperativo riguarda la responsabilizzazione delle comunità locali e di tutti i livelli istituzionali presenti. in modo molto puntuale, facendo affidamento anche sul percorso che ha visto in particolare in Emilia-Romagna il coinvolgimento diretto, a partire dal dal Commissario, di tutti i livelli istituzionali in una sede permanente, che in questo decreto-legge è stata individuata in quattro sedi regionali che fanno capo ai Presidenti delle Regioni con il coinvolgimento diretto

trasparenza, che viene realizzata attraverso l'uso di piattaforme informatiche per la gestione di tutte le risorse e la rendicontazione puntuale di tutti gli interventi. gli interventi. Esso si lega strettamente al quarto, relativo alla legalità ed al contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata attraverso la creazione di meccanismi di selezione e di controllo delle imprese incaricate incaricate dei lavori e l'individuazione, presso il Ministero dell'Interno, di un ufficio speciale in grado di coordinare tutte le Forze dell'ordine e tutte le istituzioni attraverso una condivisione delle informazioni e delle banche dati per rendere più snello il lavoro di verifica, di selezione e di controllo, a partire dall'onorabilità delle imprese che dovranno agire in questo territorio. Infatti, come sappiamo, laddove ci sono molte risorse pubbliche, l'interesse delle organizzazioni criminali aumenta come anche la loro capacità di adattarsi alle norme, di aggirarle e costruire modalità di inserimento e di infiltrazione alle quali dobbiamo opporre le barriere più alte e la strumentazione normativa e culturale più avanzata possibile.

che i loro uffici e le loro imprese hanno subito. Ovviamente, oltre a questo, ci sono i risarcimenti per tutto ciò che è patrimonio pubblico essere di grande pregio, soprattutto dal punto di vista culturale, in un territorio che ha fatto delle eccellenze ambientali e culturali un motivo di vanto e di promozione di un settore importante come quello

e conservazione, che è di qualità e contraddistingue le eccellenze alimentari che, unitamente alle bellezze ambientali e culturali, anche per anche per questa parte d'Italia, rappresentano il *made in Italy* nel mondo e, per questo territorio così duramente colpito, sono elemento fondamentale di futura

alcune proposte che volevo riprendere, in particolar modo quelle che si riferiscono alla disciplina del regime fiscale inerente le

settimane e mesi queste si sono prodigate, e lo stanno ancora facendo, per raccogliere risorse da mettere a disposizione di progetti specifici. e accolta in Commissione è tesa a migliorare la trasparenza e il sostegno da parte di questi soggetti alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi. Ancora, sul tema delle somme raccolte mediante donazioni, un altro emendamento a mia firma ha voluto assicurare l'impignorabilità di queste somme, in analogia a quanto si sta già facendo in altri territori, nella gestione delle contabilità straordinarie legate al potere del Commissario straordinario. Mi ha fatto molto piacere che sia stato accolto anche un emendamento che

nello stesso sito o in altri siti, perché di pregio sia per il materiale sia per la storia che si riferisce a quegli

che vieta l'installazione di *slot machine* nei territori colpiti dal sisma sino al 31 dicembre del 2017. del 2017. Proprio nei giorni immediatamente successivi alle scosse del 24 agosto, infatti, alcune imprese del settore si sono prodigate per mettere a disposizione

di queste macchinette. Abbiamo cercato di impedirlo per proteggere e mettere in condizione quelle popolazioni, che vivono una condizione di difficoltà e sicuramente hanno una maggiore disponibilità di tempo libero, di non essere condizionate da queste

di cui trattiamo in questo decreto, l'autorizzazione a cedere i beni in proprietà dello Stato, assegnati agli enti territoriali e non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali, con la possibilità di rimetterli in gioco laddove è stato dichiarato, in particolare, lo stato di emergenza e laddove sia stata appurata l'utilità di tali impieghi nell'ambito delle gestioni emergenziali. È un'altra di quelle proposte che ha provato a dare un contributo ulteriore rispetto

anche la discussione tenutasi in quest'Assemblea sulla prospettiva, che il Governo ha dato, di indicare un grande progetto di ricostruzione attraverso il simbolo di Casa Italia.

dal Governo, ora impegnato in modo stringente nel rispondere a questa emergenza. Al tempo stesso, però, l'Esecutivo ha avviato un lavoro molto importante per mettere in campo una serie di misure ed azioni di carattere preventivo finalizzate al miglioramento sismico degli edifici del nostro Paese e alla messa in sicurezza dei territori più vulnerabili. opera era già stata anticipata attraverso diversi provvedimenti, ma adesso il Governo ha dovuto sistematizzarla all'interno di un'unica progettualità che ha coinvolto tutti i soggetti portatori d'interesse del nostro Paese e che sta coinvolgendo le competenze più

il lavoro che si sta facendo sarà assolutamente coerente con questa grande progettualità che il Governo ha voluto mettere in campo. È una sfida che possiamo vincere tutti insieme unendo le migliori forze e le competenze già all'opera nelle cinque Regioni per riuscire a mettere in campo un percorso celere, efficace e anche qualitativamente alto, di ricostruzione e al tempo stesso per dare un buon esempio a tutto il Paese di come si può fare ricostruzione e mettere in sicurezza il territorio per il futuro.

tutti gli emendamenti, ovvero di buona parte di essi, attribuisce all'*iter* legislativo una velocità evidentemente finalizzata a intercettare con maggior tempestività i bisogni di queste popolazioni, che sono state pesantemente colpite da eventi sismici drammatici.

e che declina i principi del rispetto per i nostri fratelli sventurati che hanno vissuto e vivono questa situazione di difficoltà.

Tuttavia, anche a beneficio del Resoconto di Assemblea e per il valore che ha il Resoconto dei lavori parlamentari in una discussione proficua, produttiva e utile richiamo l'attenzione del Governo e del relatore su tre punti, con una valutazione molto rapida che parte dalla necessità di armonizzare il contenuto dell'articolo 5 con quello dell'articolo 14. Entrambi gli articoli si riferiscono alla ricostruzione e alle iniziative che lo Stato italiano (nella fattispecie il Governo e noi del Parlamento con il Governo) intende realizzare al fine di dare efficace e tempestiva attuazione alle attività di ricostruzione. Ebbene, per quanto attiene alle ricostruzioni di cui all'articolo 5, che si riferiscono all'ambito privato, è espressamente previsto un richiamo alle strutture sanitarie e sociosanitarie-assistenziali operanti nell'ambito privato. privato. Nell'articolo 14, invece, l'attività di ricostruzione riferita all'ambito pubblico è generica, poiché non fa un riferimento specifico a quella parte di ricostruzioni attinenti a un comparto che è particolarmente rilevante. Accanto alle scuole, che sono espressamente citate, non compare in modo puntuale e preciso (come ritengo sia invece opportuno e come

sanitarie e sociosanitarie operanti in quel territorio che evidentemente abbisognano di interventi strutturali. Questa è la prima richiesta che affido al relatore: la possibilità che all'articolo 14 venga espressamente contemplato il riferimento alla costruzione degli edifici che svolgono attività sanitaria e sociosanitaria-assistenziale. il seguente. Abbiamo necessità di capire nell'ambito della sanità come stanno le cose, quali sono i danni cagionati alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, perché soltanto attraverso un monitoraggio degli effetti (purtroppo in alcuni casi drammatici) che si sono registrati sulle strutture sanitarie, abbiamo la possibilità di comprendere qual è l'entità del danno e stanziare conseguentemente le somme. Quindi, relativamente a questo punto: monitoraggio dello stato di salute degli edifici destinati all'attività sanitaria; individuazione e valutazione economica del danno;

ad esempio, di una farmacia, vi sia la possibilità che venga espressamente prevista, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, in particolare all'articolo 5 della legge n. 362 del 1991 relativamente al decentramento, la possibilità di un trasferimento oltre i confini del Comune. In merito a questo emendamento, il Governo e il relatore hanno espresso parere contrario sostenendo che l'obiettivo del mio emendamento si pone in contrasto con la necessità di mantenere, ove sia possibile, all'interno del Comune tutti i servizi fondamentali. Non v'è dubbio che sia ragionevole e condivisibile la posizione del Governo, ma naturalmente l'emendamento da me proposto si riferisce a casi assolutamente particolari, come la presenza di un servizio di pubblica utilità quale è quello di farmacia - come

l'esercizio di farmacia possa continuare a svolgere la sua attività anche oltre quel Comune che si è depauperato di popolazione, garantendo magari alla residua, minima, popolazione rimasta nel Comune al quale ci riferiamo il servizio di farmacia attraverso l'istituzione di un dispensario. Sono i tre punti che credo sia utile utile valutare e che affido alle considerazioni e alle determinazioni che il Governo e il relatore vorranno assumere

i sindaci e gli assessori della Val Serina e di Oltre il Colle, in provincia di Bergamo, che sono presenti in tribuna e assistono ai nostri lavori, tra i quali è presente il sindaco di Oltre il Colle, che è un nostro ex collega, il senatore Carrara. *(Applausi)*.

l'attenzione alle strutture sanitarie e, in generale, al ruolo del sistema sanitario in un momento di grande difficoltà come quello delle catastrofi. dal semplice fatto che purtroppo questo provvedimento è stato adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza il concerto con il Ministro della salute. Il Ministero della salute è assente ed è assente l'attenzione alle strutture sanitarie e alle politiche che, in condizioni di emergenza, devono essere adottate per garantire alle persone bisognose l'accesso completo alle cure. Mi permetto di sottolineare alcuni aspetti che probabilmente chi non è addetto specificamente ai lavori non conosce. Proprio nel giorno del terremoto dell'Aquila del 2009, l'Organizzazione mondiale della sanità dichiarò di dedicare la Giornata mondiale della salute

Infatti, come giustamente aveva precisato l'Organizzazione mondiale della sanità in quell'occasione, gli ospedali non sono strutture come tutte le altre: che, proprio in caso di catastrofi, di sisma, di situazioni di grande difficoltà, devono essere in grado di garantire l'accoglienza e l'assistenza alle persone e, quindi, devono essere più sicure - se così si può dire - di qualunque altra struttura. Altrimenti, come è successo nei territori in occasione del disastro dell'Aquila e anche recentemente, se crollano gli ospedali, le persone - e sono tante - che hanno bisogno di ricevere assistenza devono essere trasferite lontano e, quindi, le difficoltà sono ancora maggiori. Ebbene, mi permetto di chiedervi di prestare due minuti di attenzione, perché questo Paese non può continuare a dimenticare il problema della sicurezza delle strutture sanitarie nelle zone a rischio di catastrofi naturali. *(Applausi della normativa disattesa da tempo dai livelli centrali e regionali. C'è un'ordinanza del Presidente del Consiglio del 2003 che stabiliva che, entro cinque anni, e quindi entro il 2008, bisognava procedere alla valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità della Protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Ieri ho molto apprezzato l'emendamento 14.0.1 che è stato approvato dalla Commissione bilancio, a prima firma del senatore Mandelli (che ho sottoscritto), che chiede che questo processo

2. Proprio per questo ritengo che la dimenticanza delle politiche per la salute e la mancanza del Ministro della salute, nell'ambito del provvedimento di cui ci stiamo occupando, sia grave. Ed è grave soprattutto il fatto che all'articolo 14 - come hanno già detto altri colleghi - non si parli espressamente

essere oggetto di attenzione per la ristrutturazione pubblica, delle strutture ospedaliere e delle restanti strutture sanitarie e sociosanitarie. Chiediamo che tutto ciò venga inserito espressamente, perché si ponga

ha dato assoluta contezza dei contenuti del decreto-legge. Prova ne è il fatto che, sia per questo motivo ma anche per il senso di responsabilità dell'intero Parlamento, oggi si sta arrivando a un sostanziale ritiro

Questo lo dico ovviamente perché anche io vengo da una zona che ha vissuto una tragedia similare, 50 anni fa (48 anni fa), e ne ho ancora piena e viva la memoria, allorquando, il 14 e il 15 gennaio 1968, circa 30-40 paesi della Sicilia vennero devastati in maniera irreversibile.

e com'era e di non disperdere non soltanto i beni storici e monumentali, ma soprattutto l'identità culturale e quella sorta di stratificazione sociale e sociologica che ha tenuto unite, nel corso dei secoli e dei millenni, le popolazioni dell'Appennino. Non voglio dilungarmi nell'illustrare il provvedimento.

n. 205 del 2016, che certamente integra e migliora il provvedimento sul terremoto. È questa un'altra occasione perduta per affrontare una calamità naturale drammatica,

Ci vorranno anni per cancellare dalla mente e dal cuore delle popolazioni delle Marche, dell'Umbria, del Lazio e dell'Abruzzo il terrore che tali eventi hanno procurato a centinaia di migliaia di persone. Non si può affrontare in questo modo una tragedia così grande. Il provvedimento in esame è illeggibile, renderà lunga, difficile, perigliosa e complicata la ricostruzione. Sono già trascorsi tre mesi dal primo evento ed è ancora tutto fermo: siamo ancora al punto zero. Siamo di fronte a un articolato illeggibile, ridondante, eccessivo, basato sulla sfiducia, sulla diffidenza e sulla cultura del sospetto. Innanzitutto, non si può procedere speditamente con una quantità di strutture

Che grande confusione! È possibile che non si possa fare un protocollo chiaro, che sia comprensibile al cittadino per poter accedere alle risorse previste dal provvedimento? Temo che la ricostruzione durerà come quella del Belice. Con questo provvedimento avete dato l'immagine di un Paese allo sfascio, nel quale non ci si può fidare di nessuno, né dei cittadini, né delle imprese, né dei professionisti. È il Paese che avete realizzato negli ultimi venti anni. Da cinque anni governate in maniera indiscussa e incontrastata il Paese: gestite lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le municipalizzate, le partecipate. Siete voi che gestite tutti gli appalti nel Paese. Avete nominato un commissario straordinario perché non vi fidate dei vostri Presidenti di Regione, tutti e quattro del PD, altrimenti non si capisce la ragione per cui lo avete fatto, visto che negli visto che negli ultimi trent'anni i Presidenti di Regione hanno gestito tutte le calamità naturali avvenute nel Paese. Non siamo contro Errani, che è una persona certamente autorevole e competente, ma non capiamo l'esautorazione e la mortificazione dei Presidenti di Regione, che conoscono bene il territorio e che in questo momento non hanno altro da fare, perché ormai le Regioni sono ridotte ad aziende sanitarie e hanno poco da legiferare; basta guardare agli ordini del giorno dei Consigli regionali. Avete inventato un'altra centrale unica di committenza, perché non vi fidate di quelle provinciali che già sono operanti. Non vi fidate dell'ANAC, perché avete istituito un'apposita struttura di missione presso il Ministero dell'interno,

Non vi fidate delle imprese, perché volete istituire una *white list* per gli operatori economici interessati a partecipare a qualsiasi attività e intervento di ricostruzione pubblica e privata; ma se una ditta non opera correttamente va radiata da qualunque albo e non deve fare né un lavoro pubblico, né un lavoro privato: una ditta di mascalzoni deve smettere di lavorare. Non vi fidate dei professionisti iscritti agli albi professionali, perché volete istituire un elenco speciale di professionisti, adottato dal commissario per la ricostruzione dopo apposito bando pubblico.

Non vi fidate dei sindaci. A voi interessa solo far credere ai cittadini che tutto è a posto e che con voi è assicurata la legalità. Volete illudere che tutto sarà ricostruito e tutto sarà risarcito. In realtà, sapete bene che non sarà così. Vi avevamo chiesto, attraverso una serie di emendamenti, di migliorare il provvedimento facendo scelte più opportune e adeguate. Non avete voluto sentire ragioni. le risorse, la Protezione civile ha stimato che per il terremoto di Amatrice si sono verificati danni per 7 miliardi di euro, mentre con le scosse del 26 e 30 ottobre, data la rilevanza e l'estensione territoriale, complessivamente sarà necessario sei o sette volte tanto. Questo evento calamitoso costerà almeno 50 miliardi e voi pensate di fare la ricostruzione con 1,5 miliardi?

Nella sostanza, le risorse che avete stanziato sono risibili rispetto al danno da riparare e agli annunci del Presidente del Consiglio di risarcire tutti i danni. Con quali risorse? Con quelle previste? Poi c'è il problema del cratere: avete individuato un cratere che presenta gravi lacune e ingiustizie. Molti Comuni, pur avendo subito danni, sono rimasti fuori dal cratere. Abbiamo il fondato sospetto che avete fatto delle scelte sulla base di ragioni politiche, anziché su criteri chiari e oggettivi. Vi abbiamo fatto una proposta rivoluzionaria, straordinaria. Vi abbiamo suggerito, per far fronte all'emergenza abitativa, di acquisire in affitto o di comprare migliaia di immobili agibili presenti sul territorio colpito dalla crisi sismica prima di consumare altro suolo, fare altra urbanizzazione e comprare casette e *box* di legno. Avete detto di no. È evidente. Avete già ordinato senza gara

Il Consorzio nazionale servizi di Bologna si è aggiudicato un bando di gara di 1,2 miliardi per la fornitura e la posa in opera di 18.000 moduli abitativi. Il Consorzio nazionale servizi e Manutencoop sono già stati sanzionati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con una multa complessiva di 110 milioni di euro

Vi abbiamo chiesto di considerare i professionisti che hanno perso studi e clienti mentre mantengono i costi di esercizio, per i quali non bastano certamente i 5.000 euro *una* *tantum* previsti perché ci vorranno anni per tornare alla normalità. Mi sono limitato a questi elementi per esprimere un parere assolutamente contrario sul

Rivolgiamo un saluto agli allievi e ai docenti dell'Istituto comprensivo «Sinopoli Ferrini» di Roma che assistono oggi ai nostri lavori. Benvenuti in Senato.

unitario di impegno registrato nel Paese. Credo che tutti noi, dopo lo scoramento, la preoccupazione e la paura

stata esaltata la capacità degli italiani a stare insieme e a rispondere alle emergenze e tragedie dimostrando un grande senso di appartenenza, di partecipazione e d'impegno;

far sì che il numero delle vittime fosse il minore possibile e che i feriti fossero ricoverati e curati.

è successo esattamente l'opposto. Abbiamo dimostrato che lo Stato c'è, è efficiente e interviene, come comprovato anche in occasione di precedenti accadimenti

quelle realtà, sono il simbolo dell'identità comunale e debbono rimanere tali, con il loro patrimonio artistico e architettonico.

illustrato dal nostro collega, il maestro Renzo Piano. Mi riferisco al progetto di Casa Italia, un intervento che deve impegnare una generazione per mettere in sicurezza tutta la dorsale appenninica, tutti i centri storici dei Comuni che si trovano all'interno delle zone ad alto rischio sismico: un intervento importante che deve avere un impegno forte da parte dell'Unione europea. Credo abbia fatto molto bene Renzi a porre la questione anche all'interno del disegno di legge di bilancio come discriminante. Non possiamo continuare a finanziare un'Europa che poi non pensa ai ai terremoti, alle scuole che in Italia sono a rischio sismico. Quelle risorse devono servire al grande piano di prevenzione Casa Italia, all'intervento che dobbiamo fare nel nostro Paese.

terremoto dell'Emilia, dove era commissario in quanto Presidente della Regione. In secondo luogo, era sbagliato, per un sisma che coinvolge quattro Regioni, nominare commissari i quattro

che dobbiamo portare avanti interventi di lunga lena e concludo ricordando una questione che è stata posta da me e da altri senatori del Lazio rispetto alla

la vecchia consolare Salaria che i romani utilizzavano per andare a prendere il sale e portarlo a Roma dall'Adriatico. Questa strada ancora percorre, grosso modo, il vecchio tracciato di epoca

da parte del Governo per ristrutturare, mettere in sicurezza e potenziare questa dorsale appenninica: no, non è stato possibile approvarlo perché esulava dalla competenza del decreto-legge ed è stato quindi trasformato in ordine del giorno. Spero che il Governo sia

sanità è giusta e ho presentato un emendamento come relatore per cogliere la necessità che venga evidenziata, anche nella ricostruzione pubblica, che pure la comprendeva, la ricostruzione degli ospedali. Sempre in tema di sanità, vorrei rispondere al collega D'Ambrosio Lettieri segnalando che la Commissione - come già detto da qualche collega intervenuto nel dibattito - ha previsto un percorso di valutazione dello stato degli ospedali in quelle zone sismiche

- deve avere particolare attenzione nei confronti dei luoghi della cultura. In particolare, voglio ricordare l'università di Camerino che è stata la più danneggiata ed è stata anche la prima a riprendere il suo lavoro ordinario, dando la sensazione di continuità della vita dei giovani

la messa in sicurezza stabile delle zone soggette a sismi e cioè le previsioni urbanistiche di strutture aggiuntive che possano consentire una salvezza costante delle persone: strutture sulle quali bisogna approfondire il tema urbanistico. Voglio dirlo perché dobbiamo puntare a un'idea di resilienza di quei territori, alla capacità di resistere alla sollecitazione continua che lì può venire. È un tema più generale dell'Italia la capacità di resistere a cambiamenti climatici, ad adattare le città e le comunità, ma in questo caso e in quei territori va pensato come resilienza resilienza alle sollecitazioni del terremoto. Ho presentato un secondo emendamento che voglio comunicare all'Aula, che è condiviso dalla Commissione bilancio e che riguarda semplicemente una correzione del personale esperto che dalla città dell'Aquila va a sostenere le pratiche di ricostruzione del terremoto dell'Italia centrale; anziché dal Comune dell'Aquila, vengono prese dal cratere. Si tratta di dieci persone

Parlamento e della politica è un segnale di speranza a tutte le popolazioni. ringrazio innanzitutto il relatore. La mia replica sarà breve, ma non può non partire da un atto di ringraziamento non formale, oltre che istituzionale, e quindi personale, ai membri della Commissione bilancio del Senato, al suo Presidente e ai Gruppi parlamentari che compongono questa Assemblea per la straordinaria disponibilità dimostrata nei lavori della Commissione per preparare la giornata di oggi per la prima approvazione del decreto-legge in esame, che rappresenta per il nostro Paese un punto avanzato nell'affrontare le emergenze che, purtroppo, negli ultimi sette anni, abbiamo dovuto vivere ed affrontare già per ben tre volte. Ripeto che il mio ringraziamento non è formale, perché dimostra che gli impegni verbali assunti da tutti i Gruppi sono stati poi calati nella realtà e nella concretezza di un proficuo lavoro della Commissione che oggi quest'Aula vedrà realizzarsi attraverso il voto che affronteremo tra pochi minuti. Vorrei soffermarmi su alcuni temi che sono stati correttamente ripresi dai

il secondo cratere venga istituzionalizzato con legge e non rimanga, così come era previsto nel decreto-legge n. 205, nell'ambito di un'individuazione relativa alla relazione tecnica solo per quantificazioni economiche e finanziarie. Si tratta di una scelta corretta, ad avviso del Governo, ma non rende le dimensioni del cratere inamovibili. Come accaduto - ahimè - anche negli ultimi recenti episodi di terremoto, può succedere che sono ancora in corso le verifiche sulle agibilità, sui livelli e le quantità dei danni, e soprattutto soprattutto sul numero delle persone che non potranno rientrare nelle proprie abitazioni. È quindi del tutto evidente che il processo e il percorso utilizzato finora per individuare i Comuni del cratere potranno essere rimessi in campo, così come già avvenuto, attraverso il ruolo che svolgono i vicecommissari, che sono i quattro Presidenti di Regione, ai quali è stata già demandata l'individuazione della perimetrazione del primo cratere. La seconda questione è legata alla modalità con la quale, all'interno di questo decreto, noi riconosceremo i danni ai privati, i danni ai privati, quindi alle persone con le loro abitazioni, prima e seconda casa, e anche alle attività produttive. Ci sono due aspetti che ritengo di dover focalizzare in quest'Aula in modo tale che rimangano a verbale. In primo luogo, la modalità: il credito d'imposta, con il quale noi erogheremo

capacità fiscale dei soggetti titolari del credito. Infatti, in termini fiscali, il credito verrà scontato dalle banche alle quali il contribuente

alluvionale, riforma passata in Consiglio dei ministri il 28 di luglio di quest'anno. Inoltre, credo sia importante ricordare i soggetti privati che avranno diritto a questo rimborso, perché dentro al cratere c'è la garanzia del 100 per

e anche tutte le case sparse che hanno avuto danni nel caso in cui le medesime siano affittate. Quindi solo le case nelle quali non risiede nessuno e che risultino seconde case avranno il rimborso al 50 per cento, perché tutte le altre verranno ricostruite con un onere a carico dello Stato pari al 100

Ci sono due articoli, il 24 e il 25, che - di fatto - riconoscono a tutta la platea delle attività produttive un intervento di sostegno in questa fase di produzione ed abbiamo dato la conferma ai colleghi senatori commissari che gli interventi di tipo strutturale

a giorni verranno pubblicate le ordinanze che attuano il primo decreto-legge, il n. 189, e il secondo decreto-legge con l'ampliamento del cratere.

tale misura riguarda tutti i lavoratori dipendenti. In più, abbiamo introdotto, per tutto il 2017, la cosiddetta busta paga pesante, ovvero la possibilità di non avere trattenute per i dipendenti da parte del sostituto d'imposta, con un emendamento che poi voteremo

che sono il vero fronte avanzato, sia sulla fase di emergenza, che è quella che ancora stiamo vivendo, che sulla fase della ricostruzione. E non è un caso che il combinato disposto dei due decreti, quindi il testo che andremo a votare oggi, garantisca proprio ai Comuni un forte incremento di personale, perché molti dei Comuni del cratere sono molto piccoli e avevano disponibilità di personale molto ridotta. altre misure, come il ristoro dei tagli del Fondo di solidarietà e la legge di bilancio (sulla quale ci siamo impegnati, con i senatori, ad aggiungere alcuni provvedimenti), andiamo a intervenire direttamente sulla vita dei Comuni. Per esempio, già in questo decreto-legge rinviamo ulteriormente

perché, come ci racconta l'esperienza di ricostruzione sugli altri crateri, ogni mese avremo necessità nuove su cui intervenire e perché le ricostruzioni devono essere sempre e comunque gestite e vissute sul campo

delle istituzioni, per dare una risposta a questa enorme tragedia alla quale tutti insieme, come stiamo facendo oggi, dobbiamo continuare a dare risposte giorno per giorno nella concretezza della nostra attività. *(Applausi

un'illustrazione unica per diversi ordini del giorno. Tengo particolarmente al discorso di lasciare aperta l'opportunità di un contributo anche per quegli edifici che alla valutazione

Il nostro territorio è articolato, montuoso e dispersivo, perché, come ho detto ieri, si tratta di un dramma diffuso sull'Appennino, con Comuni territorialmente anche molto mettere un impalcato i costi sono altissimi. Altrimenti, facesse lui i preventivi che poi portano le ditte! Faccio anche presente che è importante una sorveglianza e una vigilanza per come tutto sarà fatto: bene vigilare e controllare, ma occorre anche sburocratizzare e quindi dare opportunità ai liberi cittadini e ai professionisti di fare e poi vigilare con i controlli. Vi è

non avere poi più risorse per il definitivo, che invece è importante. È anche importante lasciare uno spazio per la riqualificazione di tutto quel territorio che insiste su un'area altamente sismica e oggi è danneggiato abbiamo una maggiore vulnerabilità degli edifici: non c'è, infatti, un edificio, anche nuovo, che non abbia la sua bella cartina geografica di trama. Abbiamo strade che sono diventate cartine geografiche, o due centimetri, anche nelle case agibili dove si continua a vivere. Si tratta quindi di un impegno di spesa che andrà rimodulato: i 3-4 miliardi di flessibilità implicati per il terremoto non ci sono, adesso la stima

vengono abilitate a rilasciare piani, programmi e progetti anche per strutture in cemento armato complesse o altro. Altrimenti, ci troviamo con professionisti che vanno a fare i sopralluoghi impauriti dalle ripercussioni che ci possono essere anche

del danno: tanti edifici vengono considerati inagibili quando di fatto, ad una migliore e più attenta valutazione, non lo sarebbero. Si tratta di costi che si potrebbero avviare: diamo pertanto ai Comuni la possibilità di ricontrollare e gestire il tutto. Ringrazio Ringrazio il sottosegretario De Micheli per la passione, l'impegno e la concretezza. Ringrazio tutti coloro che hanno dato un contributo e invito a far tesoro delle esperienze virtuose

non spendere di più e pentirsi domani: questo è ciò che chiedo. Ringrazio inoltre per l'inclusione del Comune di Fabriano, la mia area, ma mi auguro che si lasci uno spiraglio per inglobare nel cratere anche

che interrompono i percorsi economici e impediscono ai ragazzini di andare a scuola i sindaci, se non possono sforare il Patto di stabilità, non riescono a fare

dal letto. Ci ha salvati il fatto di essere al piano terra, in una casa per noi facile: così non è stato troppo faticoso uscire e arrivare all'auto». e arrivare all'auto». Sto parlando degli allettati, che durante il terremoto non hanno potuto salvarsi, se non pochi, che sono stati trascinati a forza dai cari che li stavano guardando. Ci sono narrazioni di madri che, non potendo salvare i propri figli, si sono sdraiate accanto a loro in attesa della morte. Vorrei che le madri si sdraiassero accanto ai figli in attesa di qualcuno che li salvi, di qualcuno che sappia esattamente dove sono e che possa poi, tempestivamente, prestare loro soccorso.

l'attualità, l'efficacia e l'importanza. Già in Commissione è stato svolto un lavoro che ha portato all'approvazione di ordini del giorno, compreso anche uno nostro che riguarda la riattivazione del sistema sociale di protezione per coloro che hanno disabilità. Penso anche ai centri diurni, situazioni nelle quali l'aggregazione diventa importante. Con ciò si esprime il senso di considerazione rispetto ai più deboli: pure nelle difficoltà del terremoto bisogna tener conto di queste circostanze, soprattutto per il futuro.

cratere». In questa parte del dispositivo si prevede, infatti, un monitoraggio da effettuare subito e, poiché le risorse economiche e finanziarie sono a disposizione del commissario, le possiamo limitare alle zone del cratere. Però, avendo bene inteso quali sono le volontà

Signora Presidente, il mio è un ordine del giorno molto semplice, che tende a far valutare al Governo l'opportunità di includere fra gli interventi sugli immobili che sono stati distrutti o danneggiati dal sisma anche quelli che sono volti all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili,

Non abbiamo presentato emendamenti semplicemente per fare numero, ma per dare seguito a considerazioni di merito che sono nate dal confronto con il territorio. Nonostante il buon senso che abbiamo auspicato da parte

Proponiamo allora una misura molto semplice che prevede: l'esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dallo svolgimento delle attività da impresa nella zona franca per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività; l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per il valore della produzione netta derivante dallo svolgimento delle attività, nonché l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca. signora Presidente, sono provvedimenti assolutamente aderenti a quello che il Governo ha già fatto per il terremoto dell'Emilia-Romagna. Ci chiediamo come si possa confezionare possa convertire in legge questo decreto-legge, senza inserire questo tipo di previsione, senza dare questo tipo di attuazione. Non stiamo chiedendo la luna, ma una cosa di assoluto buonsenso, che - ribadisco - proviene da un'esigenza espressa dal territorio. Il Governo potrà dire ci penserà in un futuro provvedimento, che lo vedrà dopo. Una cosa è certa, com'è stato già abbondantemente ricordato in discussione generale: quello che si fa oggi ha senso per il terremoto; quello che non viene fatto oggi dichiara l'incapacità del Governo nell'affrontare seriamente il problema della

la legislazione che si porta avanti nel Paese per quanto riguarda le ricostruzioni prevede sempre che, ad un certo punto, quando si conclude il percorso di verifica e di valutazione dei danni e quindi si riavvia la ricostruzione, venga istituita una zona franca. L'argomento è importante, ma in questo contesto il parere resterà quello espresso in Commissione,

È stato già detto - ma credo che bisogna specificarlo ancora una volta - che questo provvedimento nasce dal pieno accordo tra tutte le parti per dare più rapidamente possibile il massimo sollievo alle popolazioni. Avevamo concordato di non presentare ulteriori emendamenti, ma se la Lega fa finta di ritirarli tutti per mantenerne uno che vale più del doppio dell'intero decreto-legge è scorretto nei confronti di questo Parlamento, della Commissione, del lavoro dei colleghi, ma soprattutto riguardo alle zone terremotate, su cui vogliono speculare politicamente perché sanno che non può essere approvato! *(Applausi avremmo potuto presentare emendamenti di questo tipo; quindi, la Lega è stata profondamente scorretta anzitutto nei riguardi degli sfollati e e di chi ha estrema necessità che venga approvato questo decreto-legge! È chiaro? È inutile che pensiate di prenderci in giro; non potete andare a spendervi questo emendamento in quelle zone perché questo non è populismo: questa è proprio slealtà nei confronti dei cittadini in difficoltà. Quindi, il Movimento 5 Stelle si asterrà, e e sappiamo bene che in Senato questo vale come voto contrario. Non è questo il provvedimento in cui dovete alzare le barricate: lo dovete fare in legge di bilancio, e vedremo cosa farete in quella occasione, perché è li che si discutono i soldi veri, non qui

se noi volevamo "vendere" questo emendamento potevamo dire che anche in Commissione siamo stati l'unico Gruppo che ha presentato la questione della zona franca, uguale identica a quella della zona franca dell'Emilia. Non l'abbiamo voluto Non l'abbiamo voluto fare proprio per dare un segnale e far sì che il Governo si impegnasse, come ha dichiarato anche in Commissione, visto che questo tema è particolarmente importante e vitale. Non

i lavoratori sono contenti di poter andare ancora a lavorare. Quello era un sistema; noi l'abbiamo presentato ed è l'unico che abbiamo lasciato, senatrice Lezzi! *(Applausi

tanto perché si capisca come si è lavorato tutti affinché si arrivasse ad un voto finale che desse una risposta forte, chiara ed anche veloce alle popolazioni che aspettano assolutamente degli interventi per poter poter ripristinare, per quanto possibile, un po' di normalità (e ci auguriamo che il lavoro di tutti quanti, fatto in maniera corale, arrivi a dare questa risposta). Vorrei comunque ricordare che sulla zona franca tutte le forze hanno lavorato e presentato emendamenti, e che da parte nostra è stato presentato un ordine del giorno accolto dal Governo. Quindi il Governo si è già impegnato e siamo certi, perché è stata una questione portata avanti in Commissione, che vorrà dare risposta ed onorare questo impegno importantissimo per l'economia,

per l'approvazione del provvedimento in Assemblea. Quindi noi siamo assolutamente convinti che questa sarà la linea. Rimaniamo coerenti con quanto fatto e accordato in Commissione, con tutto il lavoro svolto, e su questo punto ci asterremo dal voto per un fatto di coerenza,

Presidente, considerata l'importanza dell'emendamento e l'aiuto concreto che esso potrebbe dare al territorio,

emendamento in sede consultiva come sarebbe stato necessario fare questa mattina quando abbiamo dato parere di nulla osta su tutti gli emendamenti,

Il mio parere in questa sede non può che essere articolato. Dal punto di vista strettamente formale, se noi facessimo

sé, dal punto di vista dell'economia del Paese, è virtuoso perché mira a mantenere delle attività economiche garantendo uno sviluppo anche ulteriore rispetto alla fase delle esenzioni fiscali, o meglio, del rinvio delle imposte,

questo emendamento meriterebbe un'attenzione molto particolare. Il clima che abbiamo vissuto in Commissione e anche in Aula è stato caratterizzato da uno sforzo da parte di tutti i Gruppi, e naturalmente il presidente Tonini ha tenuto conto di questo

Non si può qui utilizzare questo emendamento per scardinare l'ottima collaborazione che si è costruita in questi giorni a vantaggio delle popolazioni. Tutti noi abbiamo, nel cuore e nella mente, i problemi di quei cittadini e nessuno di noi vuole speculare

perché s'ha da fare; tanto è vero che tutti i Gruppi parlamentari hanno presentato emendamenti e ordini del giorno, diversamente impostati, sulla zona franca. Per esempio, io avevo presentato sia un emendamento che un ordine del giorno

afflitte da questi eventi calamitosi, per dare sostegno all'economia del luogo, si desse la possibilità di valutare liberamente per gli imprenditori un regime fiscale uguale a

se l'emendamento in oggetto diventa un ordine del giorno, allora che vengano approvati, a maggior rinforzo e impegno del Governo, tutti gli ordini del giorno che prevedevano una zona franca. Tutti gli ordini del giorno presentati su una zona franca siano assorbiti

là delle acrobazie tecniche suggerite dal senatore Azzollini, la copertura di questo emendamento è chiaramente dal 2017.

Il problema è come cercare di dare risposte vere a questo e ad altri terremoti, sapere se queste popolazioni potranno rimanere dove erano, se si potrà ricostruire un tessuto sociale ed economico e una comunità intera.

Questa storia si ripete da tempo e sembriamo non renderci conto che questo Paese balla e continuerà a ballare. Sembriamo non volerci rendere conto che o si affronta il problema globalmente, con una sorta di piano eccezionale e un piano nazionale rispetto ai problemi della sismicità di questa Nazione (che aumenterà sempre di più), o non ne usciremo fuori. Queste risposte parziali ben vengano, sappiamo tutti che servono a ben poco se non diciamo esattamente quello che vogliamo fare e quel che dovremo fare. Non è venuta mai nessuna parola in questo periodo su quello che deve affrontare questa Nazione per rendere stabili non solo le strutture sanitarie, ma tutte le strutture pubbliche e - se mi consentite - anche quelle private: questo non c'è. La vera motivazione, il vero grande dibattito, che potrebbe un clima di sicurezza per gli italiani ma anche un grande clima di investimenti seri che potrebbero portare alla ripresa dell'economia con investimenti seri e mirati, non ci sono: Noi riteniamo insufficiente quello che è stato fatto e ci asterremo rispetto al problema, perché innanzitutto mancano le risposte vere a monte. Non si dà alcuna certezza, come non la si è data in altre occasioni, che si ricreeranno le condizioni perché queste comunità continuino ad esistere, socialmente ed economicamente. Tutto questo non c'è. Ci sono questi 1,5 miliardi fra mille organismi che si rimbalzeranno come al solito le mille responsabilità o cose da fare, e italianamente perderemo tempo.

il nulla qui. Di questo quando si parla? Quando interveniamo? Cosa diciamo? È mai possibile che si continui a fingere in un momento così drammatico, che peraltro continua a ripetersi da decenni? Siamo capaci

Benedetta - per me maledetta - legge Bassanini! Voglio la responsabilità diretta del politico; basta con i poteri di questi dirigenti che fanno e disfanno come meglio ritengono. Non è possibile. Queste risposte politiche per il futuro non ci sono: non ci sono delle risposte chiare per questa gente e anche per altri terremoti; non c'è la prospettiva del popolo italiano. Questa Nazione balla e continuerà a ballare sempre più: questo è il dato reale. Cosa si propone? Il nulla, il solito pannicello caldo del momento. Non è più possibile. È arrivato in Italia il momento di dire la parola «fine» e fare tutti i seri, iniziando da me, ma innanzitutto da chi ci governa e da chi ha più responsabilità. Annunciamo pertanto il nostro voto di astensione. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, con il collega Candiani siamo andati a trovare quelle comunità di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria duramente colpite dai forti terremoti del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre, anche provate psicologicamente dall'ininterrotto sciame sismico. Quelli sono territori di montagna dove le condizioni climatiche sono pesanti già da diverse settimane. Collega Cardinali, abbiamo fatto delle visite, non delle sfilate; non avevamo giornalisti e televisioni al seguito. Siamo andati in punta di piedi, bussando prima alla porta dei sindaci; e le successive volte che ci siamo tornati l'abbiamo fatto invitati dagli stessi primi cittadini. Ci siamo mossi - io e il collega Candiani - da ex sindaci, per capire le necessità e le esigenze di quelle comunità. Pensando prioritariamente di corrispondere alle necessità di cui ci siamo fatti interpreti, in queste ultime tre settimane, in un clima di leale collaborazione, il nostro Gruppo ha

per la consegna dei decreti, ancora una volta annunciati in conferenza stampa da Renzi ma di fatto resi disponibili con diversi giorni di ritardo. I tempi per la fase emendativa purtroppo sono risultati troppo compressi. Abbiamo rinunciato, nostro malgrado, a segnalare diversi emendamenti che ritenevano importanti. Ci spiace che dei pochi emendamenti da noi segnalati, tra i diversi presentati, volti - proprio nello spirito citato ieri dalla senatrice Cardinali - a migliorare quello che c'è ed è migliorabile nel testo del decreto e, lo ribadisco, frutto di richieste pervenute dai territori colpiti, vi sia stata una bocciatura da parte di Governo e maggioranza. Certo, siamo soddisfatti che sia stato introdotto il risarcimento per le seconde case. La Lega è stata la prima e l'unica parte politica a chiedere tale previsione in occasione della riunione congiunta delle Commissioni ambiente di Camera e Senato lo scorso 1° settembre alla presenza del sottosegretario De Vincenti, all'indomani del primo terremoto di Amatrice. Non introdurre questa previsione, che ci era stata raccomandata dai sindaci di Amatrice, Accumoli e Arquata, avrebbe certamente impedito la ricostruzione di quei bellissimi borghi che nel corso degli anni hanno vissuto uno spopolamento di famiglie che hanno però mantenuto quelle abitazioni come seconde case. Ci riteniamo solo parzialmente soddisfatti per l'approvazione di alcuni nostri emendamenti,

se uno ha subito danni dal sisma. Del documento finale, frutto della fusione dei due decreti-legge, non condividiamo però diversi aspetti. Certamente sbagliato - lo ribadiamo - è l'aver blindato il cratere. I Comuni colpiti e che restano fuori sono tanti. I cittadini e le imprese di quei Comuni esclusi non godranno dei benefici fiscali: pur avendo subito danni a propria abitazione od opificio, dovranno dimostrare con perizia il nesso causa effetto. Il relatore Lai ieri, nella sua relazione, ha detto che sono cinque le caratteristiche del decreto-legge: velocità, interventi integrati, sicurezza, legalità e trasparenza. Ebbene, iniziamo subito a fare chiarezza e trasparenza sul cratere. Noi abbiamo seri dubbi che i 69 Comuni elencati dal secondo decreto-legge siano già con efficacia nel cratere e dunque stiano già beneficiando di tutte le provvidenze. Temiamo che invece debbano attendere la conversione in legge del decreto finale. In merito saremmo contenti di essere smentiti. Ci preoccupa provvedimento in esame sia figlio della legge elaborata per la ricostruzione in Emilia, per la quale lo stesso Errani, anche lì commissario straordinario, ha dovuto emanare 459 ordinanze di applicazione, l'ultima delle quali Quella legge si è dimostrata confusa e ha generato disparità di trattamento tra i cittadini che aspiravano alla ricostruzione dei loro immobili e delle loro aziende. sbagliato, dunque, non inserire nel testo l'esplicito riferimento alle pertinenze, oppure agli impianti interni ed esterni riferiti agli edifici distrutti o inagibili che dovrebbero essere rifatti i riparati

integralmente i costi di ricostruzione di un edificio con costosi interventi innovativi e di miglioria e a consentire il passaggio da una bassa ad un'alta classe energetica e poi non riconosca l'adeguamento sismico degli edifici privati con un livello di sicurezza dell'80 per cento per gli edifici strategici come scuole e ospedali. È una follia riparare gli edifici danneggiati limitandosi al coefficiente del 60 che si è dimostrato inadatto, visto che gli edifici di Spoleto e Camerino, colpiti in passato e ricostruiti con i parametri che si vogliono qui riconfermare, sono crollati lo stesso dal Gruppo LN-Aut)*. Colleghi, quelle zone del centro Italia sono classificate ad elevatissima ed elevata sismicità. Se vogliamo evitare di spendere il doppio di risorse per rifare due volte gli edifici crollati, occorre prendere opportune misure per garantirne subito la stabilità; e il coefficiente dell'80 per cento risponde a tale criterio. dobbiamo dare un nuovo ordine alle priorità di intervento da sostenere con contributi statali. Prima viene l'adeguamento antisismico, che salva

ciancia tanto del progetto Casa Italia e poi avalla queste scelte scellerate, si dimostra ancora una volta un grande parolaio. Profondamente ingiusto è poi prevedere la sola sospensione, e per un tempo limitato al settembre 2017, degli obblighi di versamento delle tasse e delle bollette. Bisognava esentarne il pagamento per tre anni e invece niente. Pertanto, famiglie e imprenditori presto si ritroveranno costretti a pagare e pure a restituire gli arretrati. Su questo aspetto Renzi doveva intraprendere un braccio di ferro con l'Europa, su questo aspetto Renzi doveva dirottare le risorse, che continua a ribadire a ribadire che per la ricostruzione non mancano, anche se, dai numeri che vediamo nel decreto-legge, sono scarse. Sbagliato l'aver voluto rinviare l'istituzione di una zona franca per agevolare fiscalmente le microimprese localizzate nei Comuni del cratere. Negare la zona franca, ma limitarsi solo a un impegno ad attivarla, e negare la *no tax area* è un grave errore; non dà prospettive, ma solo un futuro pieno di incertezze. *(Applausi dal

e di continuare ad essere sangue e ossigeno per le comunità locali, permettendo loro di sopravvivere, resistere e risorgere. Altro che speculare, cara senatrice Lezzi, la Lega Nord è l'unico partito che in Commissione ha presentato una proposta di istituzione di una zona franca. Noi ci abbiamo pensato, il Movimento 5 Stelle no. Punto. Il Gruppo della Lega Nord, per le considerazioni sopra esposte, dunque dare un voto a favore del provvedimento. Il nostro voto si limiterà all'astensione. Non è un affronto a coloro che hanno e stanno operando nell'emergenza e nel post-emergenza, come i Vigili del fuoco, la Protezione civile, le Forze dell'ordine, la Croce rossa italiana, 1'ANPAS e le diverse associazioni di volontariato, che continuiamo a ringraziare per quanto fatto. Non è uno schiaffo alle popolazioni colpite, che continueremo, come Lega Nord, a seguire, ma ne interpreta il malcontento, che da quelle parti sta sempre più emergendo.

abbiamo orientato la nostra bussola decisamente all'interesse immediato delle popolazioni che sono state colpite dal sisma. Abbiamo orientato la nostra attività parlamentare, la nostra capacità di suggerire miglioramenti al testo e la nostra di rendere il provvedimento quanto più vicino possibile all'immediatezza dei problemi. Preannuncio il voto favorevole del Gruppo che rappresento ed è un voto favorevole espresso in occasione di un evento assolutamente straordinario. Pertanto, anche l'intervento legislativo che oggi si pone alla nostra attenzione non può che essere caratterizzato da questa straordinarietà. Ci sono stati e ci sono ancora, nel provvedimento che andremo ad approvare oggi, degli aspetti che sicuramente possono essere migliorati e che possono che possono trovare in noi una certa perplessità, per il fatto di non aver raggiunto quel livello ottimale che avremmo voluto, sempre nell'interesse delle popolazioni.

conoscere divisioni. Dovremmo infatti riuscire a mettere un attimo da parte la sottolineatura rispetto alle debolezze di un'eventuale impalcatura,

poter dare alle popolazioni colpite, ma anche a chi ci guarda al di fuori dei confini del nostro Paese, la rappresentazione di un popolo capace di stringersi intorno ai bisogni dando risposte più aderenti possibili.

Oggi dovrebbe essere il giorno in cui approviamo i provvedimenti d'urgenza per dare ristoro immediato alle popolazioni colpite e anche quello con in cui prendiamo atto e riflettiamo su quante volte siamo chiamati ad intervenire su questioni emergenziali.

che vanno dalle alluvioni fino ai terremoti, per passare alle situazioni più disparate, in cui il danno si è notevolmente amplificato per la mancanza di prevenzione

oggi vi chiediamo una cosa sola, cioè di sentirvi, come Governo, responsabili di un voto ampiamente unanime. Sentitevi addosso la responsabilità e il peso di un Parlamento che si trova unito,

regolare procedura di gara. Ci rendiamo conto che le procedure non possono che essere di urgenza, perché l'urgenza è un elemento essenziale di questo provvedimento, ma vi preghiamo: non fateci vivere l'imbarazzo di azioni e attività che siano meno che trasparenti.

l'assunzione di una responsabilità piena per una ricostruzione che sia trasparente e tenga conto del grande afflato che il popolo italiano ha dimostrato in questa vicenda.

Signor Presidente, credo che lo spirito che dovrebbe animare - e in parte ha animato - il dibattito sul decreto *post* terremoto debba essere quello di un patto per la ricostruzione e per la messa in sicurezza del territorio nazionale. Quindi, credo che le polemiche debbano restare ampiamente fuori da questo dibattito. Il decreto unificato - chiamiamolo così contiene misure assolutamente indispensabili per fronteggiare un'emergenza dilatata nel tempo dal susseguirsi degli eventi sismici nel Centro Italia: Italia: deroga al blocco del *turnover* per assumere personale in grado di compiere le verifiche tecniche e assistenza abitativa alle popolazioni colpite; più poteri ai sindaci; un'amministrazione più snella; più snella; e, ancora, più fondi per gli allevatori danneggiati per costruire stalle provvisorie e moduli abitativi che gli consentano di restare nella loro terra e vicini all'azienda. L'elenco delle verifiche tecniche ancora da fare per mettere in sicurezza immobili immobili e cittadini è drammaticamente lungo. Le richieste sono destinate a crescere. Si tratta di un lavoro immane e manca il personale per svolgerlo. Per questo era necessaria la deroga al blocco del *turnover*, per assumere tecnici in grado di svolgere queste urgenti mansioni. Renzi ha assicurato che ci sarà un maggiore coinvolgimento dei sindaci dei Comuni colpiti, che chiedono più poteri perché in questi mesi si sono scontrati con le limitazioni imposte dal primo decreto terremoto, la cui impostazione non solo tendeva a centralizzare le procedure d'intervento, ma rischiava di ostacolare, a causa delle lentezze burocratiche, il tempestivo adempimento delle attività necessarie per la messa in sicurezza delle aree danneggiate, anche e soprattutto quelle appartenenti al patrimonio culturale del Paese. Modificare il primo decreto è stato, dunque, un passo nella giusta direzione, perché, rispetto al tipo di evento per cui era stato emesso, ora ci troviamo di fronte a una situazione completamente diversa. Il decreto, in questo senso, accoglie molte delle richieste nazionale dei Comuni italiani (ANCI). In particolare, viene attribuito al Commissario straordinario per la ricostruzione il compito di integrare l'elenco dei 62 Comuni già individuati nel cratere, alla luce dei nuovi danni causati dal continuo sciame sismico e attraverso l'individuazione di criteri. Governatori e sindaci hanno chiesto meccanismi più rapidi anche per i cittadini per avere le certificazioni necessarie dai tecnici della Protezione civile, quelle che sono poi necessarie per compiere i lavori di riparazione e ottenere rimborsi e risarcimenti. Il decreto unificato è chiamato, quindi, a riparare tutte queste falle. Non è solo una questione di fondi: si tratta di ripensare la macchina organizzativa per gli interventi nelle zone colpite, a fronte di un dramma che sembra interminabile. C'è un problema di tenuta del tessuto economico, di cui dobbiamo occuparci, oltre che di primo soccorso, la sistemazione degli sfollati, la messa in sicurezza di ciò che è rimasto in piedi, la ricostruzione. L'emergenza principale di cui il decreto si occupa è proprio quella di garantire un'adeguata assistenza abitativa alle popolazioni colpite. Per fronteggiarla, si prevede che il dipartimento della Protezione civile possa, con procedure rapide e trasparenti, acquisire i *container* e, sulla base delle indicazioni dei Comuni, individuare le aree sulle quali installarli. Per favorire il rientro nelle case con danni lievi, che hanno bisogno soltanto di interventi di immediata riparazione, si prevede che i proprietari, previa presentazione di apposito progetto firmato da un professionista abilitato, possano procedere al ripristino dell'agibilità degli stabili. Si velocizzano, insomma, le procedure. Per la messa in sicurezza del patrimonio storico e artistico, inoltre, i Comuni interessati possono fare direttamente gli interventi indispensabili, dandone comunicazione al Ministero dei beni culturali. Ma il problema - credo questo sia il punto su cui concentrarci non si ferma qui; c'è un obiettivo di ben più ampio respiro da perseguire: la messa in sicurezza di un territorio a rischio sismico che copre il 60 per cento delle Regioni italiane. Il Fondo per la prevenzione sismica, approvato all'indomani del terribile terremoto de dell'Aquila, programmato su sette anni, dal 2010 al 2016, per un importo complessivo di 965 milioni di euro, si è dimostrato del tutto insufficiente, dal momento che tale somma, seppur cospicua, «rappresenta - secondo il dipartimento della Protezione civile - solo una minima percentuale, forse inferiore all'1 per cento, del fabbisogno che sarebbe necessario per il completo adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche». C'è una riflessione da fare: dal 2010 al 2016 è stata stanziata nel Fondo per la prevenzione del rischio sismico una somma inferiore a un miliardo di euro, mentre nello stesso periodo il valore degli importi detraibili per la sola riqualificazione energetica, ossia l'*ecobonus*, ha superato i 12 miliardi. Prevedere un riequilibrio che favorisca una sostanziosa detassazione degli investimenti privati nel consolidamento antisismico sarebbe un passo nella giusta direzione. Se si guarda a quanto ha speso lo Stato italiano negli ultimi cinquant'anni per le ricostruzioni dopo i tanti terremoti registrati, si evince che un grande piano di consolidamento antisismico avrebbe fatto risparmiare. Quello italiano è purtroppo un ritardo epocale. Intervenendo sempre in conseguenza delle emergenze e mai in modo strutturale per un'adeguata prevenzione, si è di fatto speso molto, ma male. Secondo una ricerca del Centro studi del consiglio nazionale degli ingegneri risalente al 2014, la somma in valori attuali dei soli interventi statali di ricostruzione realizzati dal 1968 al 2012 è stata superiore a 121 miliardi di euro; mentre un adeguamento antisismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private e delle opere infrastrutturali strategiche sarebbe costato all'incirca 100 miliardi di euro. Un coerente piano di prevenzione avrebbe dunque fatto risparmiare e al contempo salvato decine di migliaia di vite umane. Il programma Casa Italia, varato dal Governo dopo il terremoto di agosto, va finalmente nella giusta direzione. Passo all'ultimo punto. È in atto un contenzioso tra l'Italia e l'Unione europea sulle spese eccezionali sostenute per i danni del terremoto e l'accoglienza dei migranti. La richiesta di più *deficit* per questi due eventi eccezionali è sacrosanta, ma l'Europa, ancora una volta, nicchia. Eppure esiste il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, varato nel 2002 e da allora utilizzato per 72 interventi in 24 Paesi per concorrere alle spese connesse a catastrofi naturali, con un'erogazione totale di quasi 4 miliardi di euro. La struttura del Fondo è buona, ma le sue possibilità di intervento sono limitate a soli 500 milioni di euro annui. Esso potrebbe essere potenziato in varie direzioni, tra cui quella della concessione di prestiti a lunga scadenza e a tassi agevolati agli Stati colpiti da calamità. Ciò richiederebbe un potenziamento del Fondo, attualmente finanziato sul bilancio europeo, il quale, insieme alla concessione di maggiore flessibilità sul *deficit*, potrebbe venire incontro alle esigenze di un Paese come il nostro, che sta fronteggiando due emergenze assolutamente eccezionali.

non solo per senso di responsabilità, ma anche per dare il segnale di un valore politico nuovo nuovo su una questione così drammatica come quella degli eventi sismici di questi ultimi mesi.

abbiamo fatto un ottimo lavoro dal punto di vista emendativo, tra l'altro componendo

delle condizioni di vita sociale nelle zone colpite. Mi preme intervenire su un aspetto

collegando gli interventi di soccorso e prima messa in sicurezza con le prospettive di ricostruzione.

potenziando la figura del Commissario e superando la concezione del Commissario quale espressione diretta delle amministrazioni locali, individuando una persona che abbia maturato già esperienze e competenza professionale su questo argomento e mettendolo in relazione positiva con il capo del dipartimento della Protezione civile, che bene ha operato e opera in queste circostanze. Penso che questo sia l'embrione normativo su cui si può lavorare per arrivare finalmente - lo ripeto al Governo perché glielo abbiamo detto tante volte e penso che il Governo non si sia dedicato abbastanza - alla predisposizione di una legge quadro sulle calamità naturali e sugli eventi sismici, che consenta già di avere un'impalcatura normativa in grado di attivare ogni livello di intervento destinato alle zone colpite. È necessario farlo in maniera tale che il tempo che si utilizza, soprattutto a ridosso dell'evento calamitoso e della situazione tragica, sia ridotto

che ancora non si è ripreso, che non ha avuto le stesse provvidenze che hanno avuto altre aree del Paese interessate da eventi calamitosi. necessario che ci sia equità in questi interventi, che non si facciano differenze, che non vi siano situazioni privilegiate e altre dimenticate, e per fare questo c'è bisogno di una legge quadro, non di un decreto-legge *ad hoc* per ogni alluvione, incendio o terremoto.

per questioni di territorio, di condizione dei suoli, di problematiche idrogeologiche, è soggetto a eventi di questa natura. Penso, allora, che questo sia un buon provvedimento sotto il profilo dello schema degli interventi proposti, dell'organizzazione delle autorità pubbliche, della collaborazione tra il Commissario - che ha capacità derogatorie proprie tutte indirizzate verso la qualificazione degli interventi, anche ricostruttivi, e per il superamento dell'emergenza - e il dipartimento di Protezione civile, che invece è ormai all'altezza di intervenire con prontezza in tutte le situazioni particolarmente urgenti. in questo testo ci sia una buona elaborazione normativa per quanto attiene anche all'organizzazione degli interventi utilizzando il potere di determinazione del commissario, delle ordinanze commissariali, e quindi quella elasticità e quella possibilità di adattamento a ciascuna realtà che vale la pena di considerare. Penso anche che noi dobbiamo avere un certo tipo di professionalità da incaricare per lo svolgimento delle funzioni

dopo la fase di stabilizzazione, anche per il sostegno positivo di tutta l'attività di ricostruzione e di ripristino delle condizioni originarie precedenti l'evento calamitoso, là dove possibile, come possibile e al massimo possibile.

e che non sono all'altezza, anche per le strutture di cui dispongono, di svolgere specifiche attività come quelle che sono invece riconducibili all'attività di commissario. Penso che il Governo dovrebbe utilizzare questo contesto per fare una proposta, che sia finalmente una proposta di legge-quadro, in grado di assicurare al Paese, in ogni momento,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, quando nel mese scorso abbiamo approvato la mozione su Casa Italia, c'è stato un consenso unanime nel chiedere al Governo un provvedimento rapido e tempestivo che desse risposte efficaci alle popolazioni terremotate del 24 agosto scorso. Successivamente, la grave, gravissima prosecuzione degli eventi sismici ha comportato la necessità di integrare i primi provvedimenti d'urgenza. Giungiamo oggi in Assemblea con una normativa organica che spero vivamente possa consentire alle popolazioni colpite di rialzare la testa il prima possibile. Il compito dello Stato certamente non si esaurisce con un decreto, ma è proprio da oggi che lo Stato deve continuare a far sentire la propria presenza soprattutto nella quotidianità stravolta dei terremotati. Le istituzioni devono immaginare - e lo hanno fatto in tempi rapidissimi - un percorso efficace affinché le popolazioni possano essere assistite nel migliore dei modi possibile e messe in condizioni di tornare alla normalità della vita nei rispettivi paesi in un tempo brevissimo. Bene ha fatto il Governo ad assumere decisioni tempestive nelle ore immediatamente successive a quei drammatici fatti: il 25 agosto 2016 il Consiglio dei ministri ha proclamato lo stato di emergenza giorni e ha stanziato i primi 50 milioni di euro per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Con un decreto del Ministero dell'economia è stata disposta la sospensione di tasse e tributi per i cittadini colpiti ed è stato nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione. annunciato ad inizio settembre il progetto Casa Italia, per uscire dall'emergenza sisma che attanaglia da tanto, troppo tempo il Paese. Casa Italia vuole essere una strategia complessiva, per creare le migliori condizioni di vita lavorative e per lo sviluppo del Paese. Un'azione di programmazione almeno decennale che punta a rendere organici gli interventi di qualificazione, modernizzazione e sistemazione dell'assetto del territorio. Il progetto Casa Italia dovrà permettere il coordinamento di una serie di interventi, da quelli sulle scuole, alle bonifiche, alle opere di diffusione della banda larga, alle opere contro il dissesto idrogeologico; dalla riqualificazione delle periferie alla modernizzazione degli impianti sportivi: il tutto articolato in un unico progetto complessivo che abbia linee guida chiare e una regia di insieme. Nell'ambito di questa strategia sono state adottate le prime misure e i primi stanziamenti sia con la legge di bilancio, sia con i due decreti-legge ormai unificati nella normativa che stiamo per approvare. Il decreto-legge si presenta come una normativa sistematica, che raccoglie le migliori prassi recenti, non solo relative agli interventi sismici e alla ricostruzione, ma anche alle procedure di appalto, massimizzate per trasparenza e controllo, agli interventi di sostegno economico in caso di calamità naturale, alla rinascita di territori resi fragili da crisi economiche e sociali. Il modello di intervento ricostruttivo si ispira alle migliori esperienze, mentre il modello sugli appalti assume come punto di riferimento l'esperienza di Expo Milano, con un forte ruolo di supervisione da parte dell'Autorità anticorruzione. In via generale, ai fini della ricostruzione dei beni danneggiati nel settore privato, sono erogati contributi sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti per far fronte alla ricostruzione, al ripristino o alla riparazione di edifici, attrezzature, beni mobili e scorte. Questo è un punto fondamentale. Al di là del mero contributo, la ricostruzione avverrà nei medesimi luoghi ante sisma. Questo permetterà di evitare i problemi evidenziati nelle precedenti esperienze di eventi catastrofici. Di estremo rilievo sono anche le norme relative al sostegno e al supporto della rete imprenditoriale locale, nonché quelle relative alla ripartenza delle piccole e medie industrie e al regime di aiuto per le aree industriali in crisi esteso alle aree del terremoto. Particolare attenzione è dedicata al settore agricolo, agroindustriale e turistico. Nell'intento di favorire anche la nascita - perché no - e lo sviluppo di nuove attività produttive nelle aree interessate, sono previsti finanziamenti agevolati a tasso zero per le nuove imprese e l'introduzione di ulteriori aiuti per il rilancio del sistema produttivo. In considerazione della presenza nei territori dei predetti Comuni di un elevato numero di famiglie sfollate dalle proprie abitazioni, si è inoltre reso necessario acquisire l'immediata disponibilità di *container* abitativi provvisori, in modo da evitare un prolungamento della sistemazione in tende e in altre strutture collettive allestite subito dopo i terremoti, tenuto conto dell'arrivo dell'inverno. I *container* saranno poi rimossi al cessare delle esigenze. Proprio su questo tema, è notizia di pochi giorni fa l'aggiudicazione della procedura negoziata bandita da Consip per il noleggio dei *container*. Entro dicembre, secondo la Protezione civile, la prima fornitura permetterà di assistere oltre 2000 persone nei campi che verranno attrezzati in sei Comuni che, al momento, hanno fatto richiesta dei moduli abitativi. Per la precisione si tratta dei Comuni di Norcia, Camerino, San Ginesio, Caldarola, Palmiano e chiaramente di Amatrice.

e un rapido adeguamento delle strutture esistenti, il provvedimento prevede che l'ANAS, in qualità di soggetto attuatore della Protezione civile, assuma il coordinamento complessivo degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali nazionali, regionali e locali. ANAS attua gli interventi di propria competenza e provvede direttamente, ove necessario - e credetemi le necessità sono tantissime - all'esecuzione degli interventi di competenza delle Regioni e degli enti locali in base all'effettiva capacità operativa degli enti interessati. Al fine di garantire anche in condizioni eccezionali il normale svolgimento della vita quotidiana, soprattutto per i ragazzi, per l'anno scolastico 2016/2017 i dirigenti degli uffici scolastici regionali possono derogare al numero minimo e massimo di alunni previsti per classe, di ogni ordine e grado, con riferimento agli edifici che sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici, alle strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni delle aree colpite. Il decreto legge prevede, inoltre, una serie di interventi urgenti per garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative. Nuove misure sono introdotte per garantire una maggiore tutela del patrimonio culturale, così ricco nei territori colpiti. Ad esempio, si chiarisce che, per tutti i contratti di lavoro, servizi e forniture relativi ai beni culturali, si applicano le procedure di somma urgenza. Si tratta di una scelta per omogeneizzare le procedure e guidare le amministrazioni pubbliche e gli operatori coinvolti nelle delicate operazioni di messa in sicurezza post sisma. L'azione governativa nel decreto-legge in esame non può non definirsi organica: da un lato, mira a ripristinare nel più breve tempo possibile la normalità nella quotidianità dei cittadini colpiti da sisma; dall'altro, tende a garantire una ricostruzione locale attenta e mirata a preservare o ripristinare il patrimonio artistico e culturale dei borghi fra i più belli d'Italia a dare un sostegno forte e duraturo al sistema produttivo per non disperdere il tessuto economico locale. Pertanto noi di Area Popolare voteremo convintamente a favore del decreto-legge, dando in tal modo una spinta decisiva per la rinascita dei borghi che rappresentano l'anima più profonda di un'Italia unita nel risollevarsi. Lasciatemi concludere dicendo che, come umbro, ci tengo a ringraziare tutti coloro, nessuno escluso,

Signor Presidente, i terremoti degli ultimi anni hanno portato in sé delle grandi tragedie, con un elevato numero di vittime, ma purtroppo la terra ci sta dando degli avvertimenti. In Italia i geologi si aspettano terremoti con energia trenta volte più forte di quella di Amatrice. Non si può sapere quando, né dove di preciso, ma di sicuro avverranno. A fronte di queste evenienze «bisogna essere preparati adeguatamente in termini di qualità dell'edificato». Ma in Italia si perde facilmente la memoria e manca la cultura della manutenzione che sarebbe, invece, ragionevole e di buon senso. l'inadeguatezza del patrimonio esistente e la mancanza di investimenti per la messa in sicurezza di edifici pubblici e privati sono, infatti, emerse in tutta la loro drammaticità. Intervenire significa prendersi carico dell'emergenza sì,

ma anche a quelli pubblici, fra i quali rientra tutto il patrimonio artistico, architettonico e culturale che costituisce il cuore pulsante dell'economia di quei territori. Spetta a noi contribuire a salvaguardare e conservare quel patrimonio. Spetta a noi ridare un volto a quei paesi rasi al suolo, garantendo l'identità territoriale e la cultura del luogo. Ricostruire significa garantire la conservazione e la valorizzazione del tessuto socio-economico delle località colpite, ricche di storia e tradizioni locali. Ricostruire significa agire attraverso interventi generalizzati di messa in sicurezza delle infrastrutture, ma soprattutto degli abitanti; abitanti che hanno sinora dimostrato di avere un ammirevole coraggio. Sappiamo che la forza degli italiani è straordinaria e sa andare oltre alle risorse economiche che verranno stanziate sia con questo provvedimento sia con altri che dovranno venire. Saranno forza e solidarietà unite al sostegno economico, che ciascuna istituzione non dovrà fare mancare, a consentire la ripresa. Ciò che importa in questo momento è dare la possibilità ai cittadini di Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio di avere un luogo sicuro dove poter vendere i prodotti tipici locali; significa dare un luogo sicuro dove far riprendere l'attività scolastica dei bambini; significa consentire di ricevere assistenza sanitaria in sicurezza; significa permettere il transito viario attraverso infrastrutture sicure. Se è vero che tutta l'Italia ha bisogno di un piano che metta al sicuro le case degli italiani, è anche vero che questa Italia lacerata dai drammi di agosto e ottobre non può essere lasciata sola. Non può essere lasciata sola nemmeno dall'Europa: l'Europa, pertanto, non si tiri indietro. È sconcertante accorgersi come essa sia così fredda e come chieda delucidazioni sulle spese eccezionali dovute al sisma e ai migranti, senza però dare cenni di solidarietà. Le vite e la dignità umana contano più dei vincoli di bilancio. Inutile dire che la politica non può muoversi solo a seguito di eventi eccezionali come possono essere i terremoti, non può agire solo in stato di emergenza. Eppure, ormai si sa che il 75 per cento degli immobili in Italia non rispetta alcun criterio antisismico. E non rispettare le norme antisismiche significa lasciare la vita degli uomini nelle mani della natura, che non fa sconti a nessuno quando trema così impetuosamente come nei mesi scorsi. Come disse Sandro Pertini in occasione del terremoto dell'Irpinia del 1980, «il miglior modo di ricordare i morti è quello di pensare ai vivi». Per questo motivo ricostruire celermente e con efficacia, ma nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità. Non deve più succedere quello che è accaduto a L'Aquila, dove le case ricostruite dopo il terremoto del 2009 sono state progettate e costruite male e con materiali scadenti.

Purtroppo siamo di fronte a eventi spesso imprevedibili e, per questo, è importante trovare soluzioni adeguate per mettere in sicurezza il territorio prima che determinate tragedie accadano. Ormai lo sanno tutti che gran parte del territorio italiano è in situazione di estrema criticità. Non possiamo permetterci di attendere puntualmente il disastro di turno. Lo dobbiamo ai cittadini che vivono in quei luoghi. Significherebbe sradicarli dalle loro origini, imporgli una vita che non sarebbe la loro. Ha più senso investire i soldi in prevenzione, anziché attendere gli eventi catastrofici per ricostruire. Oggi più che mai siamo chiamati ad agire per la messa in sicurezza del territorio, che significa non consumo di suolo, ma indirizzare gli investimenti per la protezione di ciò che di più prezioso abbiamo. Il Movimento chiede con forza e vigore al Governo di attivarsi, affinché non solo si indaghi per capire quali siano i reali rischi di ciascun territorio, ma anche per trovare le soluzioni pratiche per contrastarli. In oggi a ciascuno di noi viene chiesto uno sforzo che va oltre le singole ideologie politiche. È il momento di essere tutti uniti di fronte a questa tragedia. È il momento della collaborazione costruttiva: siamo chiamati a farlo in nome di una visione del nostro Paese come unica comunità. E le collettività dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto e dei successivi del 26 e del 30 ottobre, giustamente, non vogliono né scuse né retoriche, ma soprattutto non vogliono, non possono e non devono più aspettare. Intervenire tempestivamente è un dovere per noi istituzioni e un diritto per i cittadini che non hanno più una casa, una scuola dove mandare i loro figli, la bottega o il capannone dove esercitavano le loro attività commerciali e lavorative. Saremo sempre e ovunque al fianco di tutti i cittadini in sofferenza economica e sociale. Per questo annuncio il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, i due decreti-legge al nostro esame mostrano, ancora una volta, quanto sia complicato il sistema normativo del nostro Paese. Ci sono voluti ben due decreti-legge, aggiunti alle disposizioni di dichiarazione di stato di emergenza e alle ordinanze della Protezione civile, per stanziare pochissime risorse per l'intervento immediato e per la ricostruzione. Dei favolosi 6 miliardi e oltre sbandierati c'è ben poca traccia, perché quella cifra viene raggiunta solo con una programmazione ultratrentennale che andrà poi verificata nei fatti. Le cose che in questo momento interessano tutti coloro che sono senza una casa sono sostanzialmente due. La prima riguarda l'oggi, cioè sapere quali risorse sono in campo per la sistemazione provvisoria; la seconda concerne il domani, cioè vedere quanti soldi veri ci sono per la ricostruzione. Le popolazioni coinvolte dal sisma chiedono di poter arrivare alla prossima estate senza subire impotenti un inverno che si annuncia rigido, ma al contempo domandano di poter mettere mano al più presto al rifacimento delle proprie case e di riprendere normalmente le proprie attività per poter tornare a vivere e ricominciare a produrre. L'esperienza del 2012, quella gestita dal commissario straordinario Errani in Emilia, ci fa registrare l'emanazione di poco meno di 500 ordinanze per applicare una legge piuttosto confusa, con disposizioni che hanno creato disparità di trattamento tra i cittadini che attendevano un contributo statale per ricostruire la propria casa e chi attendeva un contributo per riavviare la propria azienda. Quella che avrebbe dovuto essere una ricostruzione a burocrazia zero si è rivelata una macchina ad alto impatto amministrativo. Di fronte a quella esperienza, che, alla fine, comunque, ha erogato 1.189 miliardi per le residenze e 621 milioni per le residenze e 621 milioni per le aziende, era necessario semplificare ulteriormente, era necessario pensare a una norma che sburocratizzasse, anche perché il tessuto produttivo di Umbria, Marche, Abruzzo e dell'alto Lazio è costituito principalmente da aziende piccolissime, a conduzione familiare, dove al piano terreno c'è l'attività e al primo piano l'abitazione. una storia tutta italiana di produttività di altissima qualità, che va tenuta nella dovuta considerazione. Per ora le risorse sono di gran lunga inferiori a quelle annunciate e l'impatto della burocrazia che ci consegna il decreto-legge n. 189 sembra ancora più importante. E non c'è traccia di semplificazione nemmeno nelle norme aggiunte dal maxiemendamento che traspone nel primo decreto il contenuto del decreto-legge n. 205. Capiamo bene il rischio di infiltrazioni mafiose e comprendiamo la necessità di controlli, ma i tempi che annuncia il meccanismo elaborato dal decreto in esame sembrano davvero essere lunghi e macchinosi. Inoltre, se valutiamo le risorse stanziate per l'anno in corso e se aggiungiamo quelle per il prossimo anno, le somme messe in campo sono veramente poche. Infatti, il grosso delle somme destinate al terremoto sta nella legge di bilancio 2017, che è ora all'esame della Camera. Ma se si fa il saldo di quanto è contenuto nella prima sezione (la vecchia legge di stabilità) e quanto inserito nelle missioni della seconda (la vecchia legge di bilancio vera e propria), rispetto alle somme già previste a legislazione vigente non sembrano esserci somme aggiuntive. Al contrario, la missione relativa al soccorso civile, che comprende gli interventi per le calamità e i fondi per la Protezione civile, passa dai 3.227 miliardi del bilancio di assestamento 2016 ai 2.906 miliardi del 2017, e quindi con una dotazione di 320 milioni in meno. Per quanto concerne gli interventi di sostegno, attraverso il sistema della fiscalità, vi sono 100 milioni rispetto ai 431 già previsti con il sisma del 2012 per il credito di imposta, correlati ai finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata), 200 milioni sono dati per la ricostruzione pubblica, ed ecco che si arriva a 300 milioni, cioè meno dei 320 appena tagliati. A questi 300 milioni si affiancano, ma non si aggiungono, altrettanti soldi dei fondi europei, che erano comunque già nella disponibilità delle Regioni interessate. Inoltre, nel decreto in esame, che assorbe il secondo, le risorse per i contributi sociali non versati nel 2017 vengono vengono recuperate dallo Stato già nel 2018 e, quindi, si tratta solo della sospensione per un anno. Per quanto concerne i tributi non riscossi nel 2016, addirittura sono richiesti dall'Agenzia delle entrate già nell'anno 2017: anche qui un solo anno di tregua. Da notare che le uniche somme cui lo Stato rinuncia veramente sono le imposte sulla casa, per un importo prossimo ai 38 milioni annui. È davvero singolare che la rinuncia a riscuotere valga solo per i prossimi cinque anni, mentre la ricostruzione è prevista in oltre trent'anni. Ci sarebbe mancato solo che lo Stato pretendesse il versamento di IMU e TASI su case disabitate, perché crollate, lesionate o non agibili. I soldi veri rimangono quindi i 191 milioni netti del primo decreto, che vanno ad aggiungersi ai 130 milioni stanziati dalle tre ordinanze, peraltro già utilizzati per la primissima emergenza. I fondi previsti per gli interventi per la sicurezza dell'edilizia scolastica, ovvero per la protezione del suolo, sono spalmati a livello nazionale. Infatti, sono in parte spazi finanziari per Comuni e Regioni, già programmati e coperti nel bilancio precedente, che sembrano non aggiungere un centesimo alla dotazione esistente per l'anno precedente il 2017; in ogni caso, sono fondi destinati non esclusivamente Quello che però ci lascia veramente perplessi è il fatto che, mentre il Governo Renzi non riesce a trovare risorse vere per i territori terremotati, continua a reclamare in sede europea una flessibilità di bilancio per il terremoto per lo 0,2 per cento del PIL, cioè quasi 3,4 miliardi di euro. Come abbiamo visto, nemmeno la somma delle poste esistenti e delle nuove risorse finalizzate alla ricostruzione porta a questa cifra. Al contrario, ci sono risorse ingenti per l'accoglienza dei migranti, che ormai è diventato un mega *business*, considerato che per il 2017 l'Italia arriverà a spendere una cifra vicina ai 4 miliardi di euro, dopo avere speso speso 3.320 miliardi nel 2016. Qui ovviamente i soldi ci sono. Spiace fare confronti, ma è giusto che gli italiani sappiano che per ogni migrante viene spesa la cifra di euro 975 euro al mese, mentre per la sistemazione di ogni persona colpita dal sisma vengono dati 200 euro al mese, con un tetto massimo di di 600 euro a famiglia. Ci sarebbe piaciuto che il Presidente del Consiglio alzasse la voce in Europa per ottenere più risorse per gli italiani sconvolti dal terremoto e non per facilitare l'immigrazione nel nostro Paese. Ci si accorge solo ora, dopo quasi tre anni di Governo, che l'Italia è contribuente netto dell'Unione europea per 8 miliardi l'anno. Ma la richiesta di flessibilità di bilancio, di nuovo indebitamento netto, va fatta per cose concrete, affrontando, veramente, con risorse importanti, la ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio e non certamente per ingrassare le organizzazioni che si arricchiscono con l'accoglienza dei migranti. Concludendo, sono passati tre mesi dal primo terremoto e le popolazioni coinvolte nel sisma sono stremate e necessitano di aiuti. Per questo valutiamo il testo in esame come un piccolo, piccolissimo passo in avanti. Non possiamo fare a meno di evidenziare che, se il Governo avesse voluto (ma avesse voluto veramente), avrebbe potuto stanziare risorse vere e dare - allora sì - una scossa, questa volta in positivo, all'economia di quei territori piegati dai movimenti di una terra che purtroppo, ancora questa mattina, non accenna a fermarsi. Il Gruppo di Forza Italia, con grande responsabilità, ha favorito un *iter* celere del provvedimento in Commissione. Ma, alla luce di tutte le considerazioni esposte, considerando insufficienti le misure contenute nel decreto-legge,

alle popolazioni e ai territori colpiti dai terremoti del 24 agosto e poi del 26 e del 30 ottobre gli strumenti necessari per rialzarsi, non arrendersi e riconquistare il proprio futuro, perché di questo si tratta: una sfida difficilissima che noi, però, riusciremo a vincere. Voglio poi ringraziare Luigi Zanda per aver scelto di affidare la dichiarazione di voto del Partito Democratico a un senatore di uno dei Comuni del cratere, di quelle comunità dell'entroterra dell'Italia centrale lungo il crinale appenninico che lega Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, le quattro Regioni colpite, la zona nevralgica di quella spina dorsale d'Italia, per usare le parole di Renzo Piano. Alla devastazione provocata dal sisma del 24 agosto, con la distruzione di Amatrice, Arquata, Pescara del Tronto e Accumoli, con il dramma irrecuperabile di 299 vittime, ma anche con il salvataggio di 238 vite, persone estratte vive dalle macerie grazie alla prontezza e al coordinamento di Protezione civile, Vigili del fuoco, Forze dell'ordine, associazioni di volontari e al lavoro instancabile di sindaci, funzionari del governo regionale e del Governo nazionale, si sono aggiunte le scosse del 26 e, soprattutto, del 30 ottobre, la più violenta in Italia dal terremoto del 1980, con epicentro tra i Monti sibillini, quelli che Leopardi chiamava i «monti azzurri». Gli sfollati, costretti a lasciare le proprie case perché inagibili, sono oltre 21.000, di cui 15.000 nelle sole Marche. Signor Presidente, io, come altri colleghi che sono qui, nelle ore immediatamente successive al sisma ho visitato alcuni dei paesi più colpiti, ho attraversato centri storici deserti perché evacuati, divenuti zona rossa, inaccessibile; ho visitato tendoni e palestre adibiti a dormitori pubblici, a mense di fortuna, a ludoteche per i tanti bimbi. Ho assistito a una reazione di grande forza e dignità da parte di anziani e famiglie della quale è difficile essere altrettanto capaci. Molte famiglie sono state divise fisicamente dal terremoto: una parte sistemata negli alberghi vicino al mare e un'altra rimasta vicino ai luoghi colpiti. È nostro compito mettere tutti nella condizione di vivere insieme, perché tra le ferite più profonde vi è quella del disagio psicologico dovuto allo sradicamento. La stima dei danni, signor Presidente, è in continuo aggiornamento e ci parla di oltre 200.000 immobili lesionati, inagibili; più di 3.000 aziende agricole danneggiate; oltre 200 stalle inagibili; 5.000 segnalazioni al Ministero della cultura per i danni al patrimonio artistico; oltre 300 istituti scolastici

dell'ospedale di Amandola, tra le province di Ascoli e Fermo, che è l'unico presidio per una zona montana molto ampia. Nell'*escalation* tra agosto e ottobre il sisma ha ampliato enormemente, per estensione e intensità, il fronte dei danni provocati, fino a coinvolgere centinaia di Comuni. Eravamo qui, in Commissione bilancio, ed esaminavamo il decreto-legge sul primo sisma, quando la nuova scossa ha reso necessaria una successiva norma, per rispondere all'emergenza nel suo complesso e nella sua natura, che nel frattempo era mutata. E questo è quello che è avvenuto. è risultato un provvedimento di grande qualità e innovazione, che permette di affrontare ogni criticità, nessuna esclusa, perché il testo che stiamo per approvare nasce innanzitutto dall'ascolto delle esigenze delle comunità locali e delle forze sociali

una *governance* partecipata, che è uno dei punti qualificanti del decreto-legge. Quella che emerge è una normativa che mai prima d'ora era stata così efficace, innanzitutto in termini di risorse messe a disposizione. Complessivamente, per quanto riguarda l'emergenza e la ricostruzione, nel decreto-legge e nella legge di bilancio vi saranno un primo stanziamento di oltre 8 miliardi e poi strumenti per la ricostruzione e il rafforzamento del tessuto civile, sociale ed economico dei territori colpiti. È un modello di intervento che raccoglie le migliori prassi dei terremoti recenti, che guarda a una ricostruzione facendo leva su procedure di appalto imperniate innanzitutto su trasparenza e controllo, con un forte ruolo di supervisione da parte dell'autorità anticorruzione. Si tratta di una legislazione che sarà tra le più avanzate in Europa. E l'Europa dovrà fare la sua parte, contribuendo ai fondi per la ricostruzione. Emergenza e ricostruzione in questo decreto-legge stanno insieme, in un progetto complessivo che vuole evitare il rischio di frammentazione e che mette in condizione di fare presto e di fare bene, di coniugare partecipazione

del Paese e della sua identità, rappresentata da quella fascia estesa di borghi appenninici da cui trae le radici la cultura europea. Va combattuto quel rischio di desertificazione e di dispersione che già negli anni scorsi era presente in zone così fragili. Va difeso per primo il lavoro, vanno preservati la filiera di impresa e il patrimonio produttivo, va data forza a un modello artigiano che è un *unicum* al mondo, un *mix* di capitale sociale e umano che è tutt'uno con i territori e da cui nascono importantissimi distretti industriali che sono vanto del *made in Italy*. Guai a disperdere il patrimonio produttivo agricolo e zootecnico o le eccellenze

così come prevede il sostegno ai lavoratori colpiti, il contributo diretto ai lavoratori autonomi e atipici, l'integrazione salariale, la busta paga pesante (senza trattenuta) per i lavoratori dipendenti. Si tratta di un provvedimento che, per rispondere e questo è un punto decisivo - amplia il perimetro del cratere fino a comprendere 131 Comuni, che sono stati individuati dalle Regioni sulla base dell'intensità e dell'estensione dei danni. signor Presidente - e voglio dirlo con forza - che le verifiche sono ancora in corso e che siamo ancora all'inizio di un percorso. Per questo le norme sono flessibili, a maglie larghe e permetteranno ordinanze interpretative. Per questo nessuno esclude che, sulla base della verifica di agibilità e della quantificazione dei danni, i Presidenti di Regione possano proporre al commissario e al Governo l'integrazione del cratere. Anzi, sono sicuro che questo avverrà. In tutti i casi, l'obiettivo è ricostruire tutto il tessuto urbanistico e comunitario

fuori dal cratere, che sono nei centri storici, nei borghi, nelle frazioni e anche alle case sparse, se affittate. Voglio dire, signor Presidente, che la polemica sulle zone franche mi sembra propagandistica, perché le norme già adesso esistenti tolgono qualunque sono molto meglio di quelle zone franche che il Governo si è impegnato a valutare dopo la fase dell'emergenza.

che sostiene i Comuni e la cui tenuta è decisiva, con l'esclusione del pareggio di bilancio, la sospensione dei mutui e degli adempimenti finanziari, l'aumento del personale, per velocizzare il monitoraggio e anche la possibilità di utilizzare i tecnici comunali per redigere le schede di accertamento.

si basa il voto del Partito Democratico. Avremo di fronte altri mesi duri e complicati e non possiamo sbagliare nulla, per la responsabilità che abbiamo nei confronti di chi ha bisogno di risposte urgenti. L'emergenza, signor Presidente, non ha colore: di fronte all'emergenza si lavora insieme e spero ci possa essere un voto un voto unanime. Sarebbe il modo migliore per dare al nostro Paese la fiducia e la forza che merita.

purtroppo sono costretto a dichiarare il mio voto in dissenso rispetto al provvedimento in esame, per correttezza, serietà e responsabilità. per almeno tre ordini di motivi. In primo luogo, le risorse stanziate in questo provvedimento sono risibili rispetto a quelle necessarie per la ricostruzione, che grazie al provvedimento in esame sarà lunga, travagliata e accidentata. Inoltre, l'elenco dei Comuni inseriti nel cratere è largamente incompleto e discriminatorio nei confronti di alcuni Comuni fortemente danneggiati, ma esclusi solo per ragioni politiche, mentre la scelta sarebbe dovuta avvenire sulla base di criteri oggettivi, in base al danno. Infine, è stata rifiutata la proposta molto sensata di acquisire parte del patrimonio edilizio disponibile sul territorio, per far fronte alle esigenze abitative, perché il Governo deve collocare i moduli abitativi già acquistati dal Consorzio nazionale servizi di Bologna al prezzo di un miliardo e 200 milioni di euro, con una scelta che determina un enorme spreco di denaro pubblico, che necessiterà di utilizzare altro suolo e realizzare ulteriori urbanizzazioni.

naturalmente compatibilmente con la ristrettezza dei tempi dettati dal calendario deciso dall'Assemblea. Tale ristrettezza dei tempi non ha consentito di votare di votare gli emendamenti e in particolare di votare il mandato al relatore. Sono stati presi in esame alcuni temi, d'accordo con i Gruppi,

del quale sia io che il collega Marino ci siamo fatti garanti per quanto sta nelle nostre possibilità - che alcuni di questi temi possano essere presi in considerazione nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio. comunque sotto gli occhi dell'Assemblea che il decreto-legge fiscale costituisce una parte importante, significativa dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, della manovra di bilancio e che il Senato non ha potuto prenderlo in esame con l'accuratezza e anche la disponibilità di tempi che sarebbero state necessarie. Credo, quindi, sia quanto mai opportuno che nel prosieguo dei nostri lavori, quando entreremo nella sessione di bilancio, questo elemento venga tenuto presente anche dal Governo, al quale mi permetto di sottoporlo possa esserci uno spazio congruo affinché questi aspetti e questi temi, che certamente interagiscono con la legge di bilancio, possano essere oggetto di una discussione ed eventualmente anche di un pronunciamento dei senatori in Commissione bilancio e poi in Assemblea. Quindi, per quanto riguarda il prosieguo dei nostri lavori, i lavori delle Commissioni riunite si sono conclusi senza un mandato al relatore ma con l'accoglimento,

recante disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. Come si desume dal titolo e dal preambolo, il decreto-legge in esame troverebbe i suoi presupposti nella straordinaria necessità e urgenza per le esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente e per ottimizzare l'attività di riscossione. Tuttavia, buona parte delle disposizioni in esso contenute (ed in particolare gli articoli l, 3 e 5) produrranno i loro effetti sostanziali solo a decorrere da giugno 2017 e oltre. Nel decreto-legge in questione, a parte le clausole di stile e le enunciazioni di principio contenute nel preambolo, non vengono elencati minimamente i fatti o le circostanze connotati dai requisiti di straordinarietà, di necessità e di urgenza che imporrebbero di provvedere con decreto-legge; requisiti che devono esservi congiuntamente tutti per legittimare l'uso di poteri straordinari, eccezionali e urgenti propri della decretazione d'urgenza da parte del Governo. Con le sentenze nn. 29 del 1995, 171 del 2007, 128 del 2008 e 22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo dell'omogeneità. Inoltre, relativamente al contesto normativo in cui il decreto-legge si inserisce, esso stride con la legge cardine in materia fiscale vigente, che è lo statuto dei diritti del contribuente, legge n. 212 del 2000, che all'articolo 4 vieta l'utilizzo del decreto-legge in materia tributaria. Si configura, pertanto, un abuso del ricorso alla decretazione d'urgenza che, nella fattispecie, rappresenta soltanto il mezzo per svilire il dibattito e l'esame parlamentare e per far credere nell'illusione di avere realizzato, con immediatezza, determinati obiettivi. Nel merito delle singole disposizioni, quanto alla prevista soppressione di Equitalia, si evidenzia che la misura si traduce, in sostanza, in un mero cambio di veste del soggetto preposto alla riscossione. Sul punto, già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 480 del 30 dicembre 1993, aveva stabilito il principio del necessario rapporto in termini di congruità e ragionevolezza tra la misura dell'aggio e la soglia di copertura del costo della procedura. La violazione dell'articolo 3 della Costituzione emerge anche in relazione alle disposizioni in materia di volontaria collaborazione per il rientro dei capitali dell'estero. Si prevede infatti la riapertura dei termini di accesso alla volontaria collaborazione, consentendo la presentazione dell'istanza fino al 31 luglio 2017 per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016. Tuttavia, la riapertura del termine di presentazione dell'istanza di adesione alla *voluntary disclosure*, non risulta accompagnata da una maggiorazione della sanzione, di fatto generando una disparità di trattamento tra cittadini rispetto alla propria posizione con il fisco italiano. L'incostituzionalità per difetto di ragionevolezza e uguaglianza, riguarda altresì le disposizioni relative alla definizione agevolata di cui all'articolo 6. La misura, che alcuni osservatori hanno indicato avere connotati «condonistici» in senso lato in sostanza, non distingue affatto tra coloro che hanno omesso di dichiarare e versare importi al fisco al solo fine di evadere le imposte (con sanzioni a carico per omessa o fraudolenta dichiarazione) e quanti, invece, hanno omesso o ritardato il versamento, non avendo la possibilità e i mezzi per farvi fronte. Significativa è poi la previsione relativa ai soggetti che accedono alla definizione avendo già in corso una rateazione: anche in tal caso, si favorisce chi aveva deciso di non provvedere in alcun modo al pagamento pagamento (con l'abbuono integrale delle sanzioni) rispetto a chi, pur avendo in corso regolari pagamenti, viene ammesso alla definizione senza il rimborso delle sanzioni già pagate. Si tratta di una evidente ingiustificata disparità di trattamento che riversa tutti i suoi effetti sulla legittimità costituzionale della norma in esame in relazione all'articolo 3 della Costituzione. Sempre in riferimento alle disposizioni in materia di definizione agevolata, si osserva infine che il ricorso alla riduzione o esclusione delle sanzioni come strumento di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive far fronte a spese dello Stato, implica un utilizzo distorto dello strumento sanzionatorio dal momento che prevale, rispetto alla funzione punitiva, la finalità impositiva. Pertanto, il prelievo derivante da tali misure deve essere assimilato a quello propriamente fiscale con la conseguente verifica di compatibilità con l'articolo 53 della Costituzione. Con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 9 del decreto-legge, non può che stigmatizzarsi l'ennesimo erroneo utilizzo della decretazione d'urgenza, peraltro sul punto palesemente eterogeneo, in tema di partecipazione italiana alla missioni internazionali di pace. Più nel dettaglio, dopo decenni di sistematiche e contraddittorie decretazioni d'urgenza, con cadenza annuale (quando non semestrale o addirittura trimestrale), al fine di garantire la partecipazione italiana alle suddette missioni internazionali, il citato articolo 9 dispone nuovamente sul medesimo ambito in modi e forme non previsti dalla legislazione quadro vigente. Ciò avviene nonostante l'entrata in vigore della legge n. 145 del 21 luglio 2016 (cosiddetta legge quadro per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali). Deve inoltre rilevarsi il contrasto tra il medesimo articolo 9 e la risoluzione n. 2240 del 2015 delle Nazione Unite, la quale non solo non contiene l'autorizzazione a passare alla fase seconda dell'operazione EUNAVFOR Med Sophia, ma esclude ogni tipo di presenza di truppe straniere in territorio libico. Alla luce di ciò, la disposizione presenta profili di contrasto con gli impegni internazionali assunti - e pertanto pienamente vigenti nel nostro ordinamento - ai sensi degli articoli 10 e 11 della Carta costituzionale. Infine, contraddittoriamente rispetto all'auspicata semplificazione, il decreto-legge contribuisce a complicare ulteriormente il funzionamento del sistema fiscale, arricchendolo di ulteriori tasselli burocratici, nuovi ed onerosi adempimenti e difficoltà ulteriori per gli operatori e i professionisti che rendono i dati disponibili ed intellegibili per l'amministrazione finanziaria. Peraltro, proprio il continuo cambiamento delle regole, oltre alle disposizioni premiali discriminatorie sopra ricordate, contribuisce a vanificare qualunque proclama di lotta seria all'evasione fiscale, laddove il citato articolo 53 della Costituzione richiederebbe interventi di tenore molto diverso da quelli adottati negli ultimi anni.

avendo avuto così poco tempo, anche in Commissione, per esaminare questo provvedimento, provo un certo imbarazzo ad ascoltare i commenti fatti a proposito dei suoi contenuti. Come abbiamo visto anche alla Camera, questo decreto-legge (e sottolineo che si tratta di un decreto-legge) contiene, come dice il titolo, provvedimenti in materia fiscale e provvedimenti definiti, definiti, da una espressione abbastanza oscura, esigenze indifferibili. Anche in questo caso, purtroppo, ci troviamo di fronte a dei titoli il cui contenuto risulta molto diverso. In questo caso, signora Presidente, colleghi, ci troviamo a dovere esaminare la costituzionalità del provvedimento che ci viene sottoposto velocemente, con tempi super contingentati, dopo che in Commissione, come ci ha detto il presidente Tonini, Tonini, è stato eiettato verso l'Aula addirittura senza il relatore. Noi dobbiamo dare un giudizio di costituzionalità su di un contenitore, che porta

per il nostro obbligo di filtro costituzionale, fermare questo provvedimento, di cui ognuno di noi, ancora una volta, deve assumersi la responsabilità e i cui requisiti di necessità e urgenza, come vedremo, nella più parte delle disposizioni in esso contenute semplicemente non esistono. L'articolo 1 reca la trasformazione di Equitalia da società per azioni (pur se partecipata pubblica) in ente pubblico economico, quando noi sappiamo che, alla conclusione dell'esercizio finanziario 2016, non esisteva alcuna necessità per questa accelerazione.

la società per azioni Equitalia in ente pubblico economico operando un doppio spregio alla Costituzione, inserendola su di una locomotiva che nulla ha di necessario ed urgente ma che è profondamente eterogenea e disomogenea.

cui, ahimè, noi dell'opposizione ci siamo ormai stancati di parlare, citando inutilmente sentenze della Corte costituzionale che ci dicono semplicemente che non dobbiamo Governo non può utilizzare il decreto-legge in maniera impropria, contraria alla Costituzione, e che noi non lo dovremmo legittimare. Oltre a questo, esiste anche l'aggravante di una violazione dell'articolo 97 della Costituzione, per cui tutti i dipendenti che operano all'interno del pubblico impiego lo debbano fare attraverso una procedura ad evidenza pubblica e ciò non accadrà per gli 8.000 dipendenti di Equitalia. Ricordiamo tutti cosa ha detto il Presidente del Consiglio, ovviamente in televisione, esistendo ormai un'occupazione *manu militari* degli spazi informativi di ogni genere (spazi televisivi, radiofonici, giornalistici): ormai siamo invasi da questa infinita campagna elettorale che ci sottopone a uno *stalking* comunicativo continuo.

in totale spregio a chi ha fatto un concorso, che non è solamente una selezione, ma una valutazione comparativa per esami e per titoli, dove esistono altri candidati oltre ai soggetti che devono essere legittimati e selezionati. e selezionati. Signora Presidente, colleghi, noi lo abbiamo fatto presente ovunque: lo abbiamo detto alla Camera dei deputati, dove naturalmente il provvedimento è passato con altrettanta velocità, perché sappiamo che purtroppo il treno di questi decreti-legge non ferma più a certe stazioni dove invece dovrebbe fermare per espressa previsione della Costituzione lo ribadisco ancora una volta. Noi abbiamo cercato di dire più volte che quando si fanno i titoli, quando si mettono i temi, bisogna fare conseguenti svolgimenti: qui qui non possiamo lavorare con le *slide*, con i proclami, non possiamo fare propaganda, noi siamo dei legislatori e ai titoli debbono corrispondere dei contenuti! Quando si parla di rottamazione delle cartelle esattoriali - e questo è un tema che tocca molto da vicino noi di Forza Italia - si deve veramente inserire sotto questo titolo un contenuto adeguato ad assistere persone contribuenti in gravi difficoltà economiche, siano esse risalenti o momentanee. fine mese si trovano nella drammatica situazione di dover decidere se pagare gli stipendi ai dipendenti, se pagare tasse, mutui, rate sui capannoni o sulle case o se pagare le imposte. Noi abbiamo presentato un disegno di legge per una rottamazione vera delle cartelle esattoriali, che non è una sanatoria, ma dà la possibilità al contribuente ottemperante, che dichiara fino all'ultimo euro ma temporaneamente non ha il

ancora una volta vuole inserire un contenuto sbagliato sotto un titolo apparentemente giusto. Non è vero che Equitalia non c'è più; non è vero che la rottamazione delle cartelle porterà benefici ai contribuenti ottemperanti. Cinque ratei di rottamazione in tempi così brevi, con la necessità di pagare il 70 per cento di quanto dovuto subito, rappresentano un vantaggio per gli evasioni fiscali e non per i contribuente E rappresentano solamente un modo per questo Governo per guadagnare presto e spendere l'ennesimo titolo in corrispondenza dell'ennesima scadenza elettorale.

Lo stesso discorso vale per la *voluntary disclosure*, ma questo è un altro tema che riguarderà un altro elemento di incostituzionalità di questo infelicissimo e arrogante decreto-legge, l'ennesimo di questo Governo. Ho parlato della parte che non avrebbe mai dovuto essere inserita in un decreto-legge ma, come tutta la materia fiscale che è destinata a regolare in maniera permanente i rapporti

a pioggia a destinatari che devono solo votare sì. Un esempio per tutti: 600 milioni alle ferrovie campane,

ancora una volta siamo costretti a porre una questione pregiudiziale sull'ennesimo decreto‑legge

per quanto riguarda questo decreto, a una violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Il primo punto è la questione della totale eterogeneità

gli insediamenti dei nomadi, a disposizioni in materia di contratti dell'ISMEA, a misure per il trasporto regionale, al finanziamento dell'attraversamento ferroviario della linea Milano-Saronno, allo stanziamento di nuove risorse per il contratto a RFI, a misure per la promozione e lo sviluppo del settore agroalimentare. E potremmo stare qui a continuare ad enumerare tutti i provvedimenti assolutamente eterogenei contenuti all'interno del decreto.

Tra l'altro Renzi si dovrebbe mettere d'accordo con se stesso, perché una volta utilizza a piene mani piccoli strumenti che possono evocare qualche beneficio

principi costituzionali che, ho ben compreso, anche alla luce della riforma costituzionale, non sono più punti di riferimento di questa maggioranza: in questo caso ci troviamo di fronte a un'operazione che, contestualmente al trasferimento della funzione di riscossione di concede una larga sanatoria prevedendo la definizione agevolata, cioè con relativa cancellazione di sanzioni e interessi, di tutti i carichi

Contrariamente a quanto si vuol far credere al contribuente, la contropartita non sarà non sarà quella di un fisco più amico, ma anzi si assisterà a un aumento della capacità informativa e della pervasività Equitalia rispetto a quella di cui disponeva in precedenza. Su questo, anche dal punto di vista delle conseguenze, forse dovremmo in qualche modo riflettere. Un'altra questione francamente incredibile, a nostro avviso anch'essa confliggente con molti principi costituzionali, è che proprio l'articolo 1, esattamente al comma 15, con riferimento all'attività di riscossione si limita a stabilire che proseguirà fino al 30 giugno

che sono effettivamente in uno stato di grave difficoltà economica, attraverso la concessione delle rateizzazioni. Il rischio molto chiaro in questo provvedimento, che vede messo in discussione l'articolo 3 della nostra Costituzione, che, da una parte, c'è una larghissima sanatoria e un regime agevolato per coloro che hanno evaso ed hanno decreti tributari molto ampi, ma hanno la possibilità di pagare, mentre, dall'altra, non vi è certezza per coloro che sono in un effettivo stato di difficoltà, per i quali non è ben chiaro se vi è una proroga delle facilitazioni. Vi è quindi una palese violazione dell'articolo 3. Per quanto riguarda, poi, il provvedimento di vero e proprio condono, perché la *voluntary* *disclosure* di fatto così

Per tutti questi chiarissimi motivi di incostituzionalità, noi riteniamo che questo provvedimento si dovrebbe fermare qui. Per questo motivo, chiediamo di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2595.

è un continuo ricorrere alla decretazione d'urgenza e infatti ci troviamo di fronte all'ennesima norma di conversione di un decreto-legge. A noi sembra che, ormai, la decretazione d'urgenza sia diventata quasi prassi in questo Paese, al punto di diventare la procedura ordinaria per la produzione di norme primarie. oltre a stravolgere tutto un sistema di pilastri normativi, essa opera il danno maggiore in una democrazia, cioè lo svuotamento del ruolo del Parlamento.

"una degenerazione in grado di oscurare principi costituzionali di rilevanza primaria" e crea, sicuramente, un problema di certezza del diritto, non soltanto perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso lo stravolgimento dell'articolo 70 della Carta costituzionale, ma anche perché (secondo danno rilevante) priva l'opposizione della facoltà di esercitare la sua stessa funzione di indirizzo e di controllo politico. Ricordiamo che l'articolo 77 della Costituzione assegna la titolarità del potere normativo in capo alle Camere collettivamente e stabilisce dei precisi limiti sostanziali (la straordinarietà e l'urgenza), oltre che formali (un'efficacia limitata nel tempo) alla potestà legislativa del Governo, la quale può essere soltanto esercitata, ma non detenuta come potere attribuito al Governo. L'eccessiva espansione del potere normativo del Governo è stata più volte censurata sia dal Capo dello Stato che da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale per l'approvazione delle leggi. Ne citiamo soltanto due: la sentenza n. che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli di un provvedimento del 2004 per mancanza dei requisiti di necessità e urgenza, e la sentenza n. 128 del 2008, che evidenzia anche la mancanza di presupposti fattuali, come la disomogeneità, che caratterizza spessissimo questi decreti-legge. Inoltre, sempre la Corte costituzionale sancisce che l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo non viene sanata dalla legge di conversione, anzi, essa è a sua volta incostituzionale per un vizio dell'intero procedimento. Ebbene, nonostante tutti questi richiami degli organi di garanzia, l'Esecutivo continua ad emanare decreti-legge: abbiamo calcolato che, mediamente, ci troviamo a convertire due decreti-legge ogni mese.

ci si "spreca" nel paventare un minimo di presupposto giuridico per giustificare il fatto che si esercita un potere non attribuito al Governo, ma alle Camere.

Secondo noi, a questo punto, l'utilizzo della decretazione d'urgenza si giustifica soltanto sotto il profilo politico: il Governo, in questo momento, preferisce adottare la decretazione d'urgenza piuttosto che fare ricorso allo strumento normale, proprio per evitare il percorso parlamentare.

contraddice anche la grande riforma costituzionale, di cui abbiamo parlato fino ad ora e su cui tra poco più di dieci giorni il popolo italiano si dovrà esprimere,

perché si sa già che verrà posta la fiducia? In meno di ventiquattr'ore il Parlamento italiano è in grado di dare il via a qualsiasi tipo di norma. Per cui gli italiani che hanno un minimo di *grano salis* capiranno che la riforma costituzionale è

Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Gaetano Salvemini-Emanuele Filiberto Duca d'Aosta» di Firenze. Benvenute e benvenuti al Senato della Repubblica.

Signora Presidente, la nostra questione pregiudiziale parte dall'analisi di quella parte del decreto-legge che è incentrata sulla riforma di Equitalia: una vera e propria riforma del sistema della riscossione,

nuovo ente pubblico economico che è l'Agenzia delle entrate-Riscossione che diventa un ente strumentale. Ebbene, proprio questo ci dovrebbe far pensare che, se fossimo in un Parlamento normale e dovessimo applicare le norme della Costituzione, così come le norme di leggi consequenziali ai principi della Costituzione, avremmo dovuto esaminare un disegno di legge di riforma della riscossione, svincolato da un decreto-legge veloce, per il quale si contingentano i tempi in Commissione e si arriverà, tra qualche minuto, al voto di fiducia. È proprio l'opposto di quello che deve fare un Parlamento, quale che sia, monocamerale o bicamerale, che normalmente deve

con una definizione agevolata delle cartelle esattoriali dal 2000 al 2016. Anche qui, ci sarebbe da discutere, ad esempio, di quali siano state o saranno le sorti di coloro che, a cavallo del 2000, erano *sub iudice*, perché magari avevano impugnato

un'operazione di "mancia elettorale", che, dagli 80 euro in poi, è una delle costanti di questo Governo. Si dovrebbe però spiegare al cittadino, possibile fruitore di quella mancia, che questo tipo di regalo ha un prezzo molto salato: la rottamazione delle cartelle genera iniquità nei confronti di quei soggetti che hanno pagato tutto per tempo e addirittura per coloro che hanno chiesto la disprezzo degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Non solo: il comma 1 dell'articolo 3 prevede la facoltà dell'Agenzia delle entrate, una

in particolare, dalla sentenza n. 220 del 2013 della Corte costituzionale, laddove si è esplicitamente affermato che il decreto-legge non può realizzare una riforma organica di sistema in ragione della natura chiaramente non

delle sorti del Fondo di previdenza per gli impiegati dell'esattoria-ricevitoria delle imposte dirette, che era a gestione autonoma all'interno dell'INPS. Nel decreto-legge non si chiariva come venivano utilizzate queste risorse; forse, con un ordine del giorno approvato in Commissione, qualche chiarimento è stato portato nelle ultime ore e questo cancellerebbe un'ulteriore perplessità. Riguardo al meccanismo introdotto dal decreto-legge per la riapertura dei termini della *voluntary disclosure*, bisogna dire che si crea un'ulteriore incertezza in merito ai saldi e alle coperture del disegno

sentito, reca interventi volti a incidere su varie materie e settori diversi dell'ordinamento. Si va dalla materia fiscale, al finanziamento degli ammortizzatori sociali, alla partecipazione di personale militari alle operazioni in Libia.

un conflitto con i principi stabiliti anche di recente dalla sentenza n. 22 del 2012 della Corte, che ha collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, richiesti dal secondo comma dell'articolo

esistono e costituiscono il presidio del fondamentale principio della separazione dei poteri e della democrazia stessa; gravi sono i profili di incostituzionalità presenti nel provvedimento

per usare un'espressione che è entrata con eleganza nella terminologia politica del nostro Paese, un'accozzaglia

In apparenza è un punto marginale, mentre in sostanza è fondamentale, perché già oggi interessa alcuni milioni di cittadini con la partita IVA, evasori da oggi fino a prova contraria. Per inciso, mi pare anche che sia il *de profundis* del fisco amico. La norma potrebbe estendersi, per come assurdamente scritta, anche ai professionisti. In ogni caso, la prospettiva è che si estenda a tutti i cittadini. Con una piccola norma viene fatto attentato a un grande principio. Si attenta al principio della libertà nell'uso della proprietà sul lato fondamentale della proprietà del denaro e, perciò, anche del risparmio. L'articolo 47 della Costituzione dispone che «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio (...); disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito». Mi pare che l'azione fatta di questi tempi da questo Governo sia un ribaltamento di questo principio. Il Governo ha cercato di tutelare il credito e lo ha fatto nel modo caotico che abbiamo visto, a partire dal *bail in* così votato anche in quest'Assemblea, su cui credo che molti tecnici, più che i politici, dovranno essere comunque assolti ma non per "non aver commesso", bensì per "non avere compreso" il fatto. In realtà qui oggi, ribaltando l'articolo 47 della Costituzione, non si tutela il risparmio disciplinando il credito, si disciplina il risparmio e lo si fa in modo inaccettabile e incostituzionale. Quella piccola norma, senza ragione e in violazione della Costituzione, introduce il principio dell'uso controllato e limitato del denaro e, perciò, del risparmio, così che le sorti del tuo denaro e del tuo risparmio vengono a dipendere dalle sorti della banca presso la quale lo «devi» lasciare. Non è che l'inizio, perché così si avvia inesorabilmente un processo che va verso il totale concentrazionario controllo della vita degli altri. È solo l'inizio. Si può dire che è solo la prima intelaiatura della gabbia prossima ventura, ma, come diceva il poeta Dante, «non t'inganni l'ampiezza de l'intrare». Può essere Può essere che il futuro sia quello della moneta elettronica, del *bill coin* e della non moneta, ma non può essere che il nostro presente sia quello della non proprietà.

dell'articolo unico del disegno di legge n. 2595, di conversione del decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 193, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. Convoco pertanto La seduta è sospesa.

La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge recante disposizioni in materia fiscale, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Per la discussione sulla fiducia, che si svolgerà entro questa sera, sono state ripartite due ore e cinque minuti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Le dichiarazioni finali di voto avranno luogo domani mattina, a partire dalle ore 9,30, e seguirà, quindi, la chiama. Dopo il voto di fiducia, l'Assemblea delibererà sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza della senatrice Bottici, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, sul disegno di legge di istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla comunità «Il Forteto».

ha preso atto della relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, e non ha fatto alcun rilievo.

posta la fiducia e quindi abbiamo evitato anche il tempo della discussione generale. Perché far parlare i senatori? Perché far dire loro le cose che non vanno? È questo che dispiace, Presidente.

Vorrei però che qualcuno mi spiegasse che cosa cambierà concretamente per i contribuenti che riceveranno le cartelle esattoriali, visto che il sistema sanzionatorio rimane esattamente lo stesso, e anzi, il profumato aggio è stato incluso tra le somme da pagare e, quindi, la definizione agevolata delle cartelle, cosiddetta rottamazione, decade. Le cartelle saranno semplicemente gestite da un ente strumentale

unico di giustizia creato appositamente al fine di accentrare e gestire le risorse provenienti dai sequestri penali amministrativi e dai procedimenti civili e fallimentari. Ricordo infatti che tali somme non sono nella disponibilità dello Stato, ma devono essere soltanto amministrate durante tutta la durata dei processi e non posso essere utilizzate se non in presenza di una sentenza passata in giudicato. Durante tutto questo tempo Equitalia incassa l'aggio, determinato annualmente con decreto del Ministero dell'economia, raggiungendo importi anche molto elevati, essendo previste procedure informatizzate e standardizzate per fare confluire al FUG denaro e titoli. Quindi, con una sola mossa, il Governo incassa, da un lato, il consenso dei cittadini cui è andato a raccontare che Equitalia non c'è più e che finalmente il renzismo li ha salvati dal mostro delle cartelle pazze. Dall'altra parte, però, cosa fa? Si tiene buona una parte dei poteri forti, salvando un importante ramo dell'ente di riscossione, che sicuramente si ricorderà del Presidente del Consiglio il 4 dicembre. Andando avanti, si abolisce lo spesometro e si rivede tutto il sistema di trasmissione dei dati, delle fatture e delle liquidazioni periodiche delle partite IVA. Così il Governo si assicura una sostanziale entrata di liquidità, pari a oltre un miliardo soltanto nel 2017, ma aggrava in maniera importante

bella riforma per sburocratizzare effettivamente il nostro sistema era forse più necessaria che non la riforma della legge costituzionale. della senatrice Fucksia).* E mentre le imprese italiane vengono sempre più aggravate, lo Stato incassa da parte sua le sanzioni che saranno immediatamente applicabili dal 2017. 2017. Non si dà neanche il tempo necessario per l'adeguamento alle società di *software house* che devono predisporre il pacchetto. Quindi, i contribuenti saranno oggetto di multe, ma a causa non di una volontaria omissione di dati, ma semplicemente di un problema tecnico.

Infine, veniamo al nodo principale del decreto-legge: la rottamazione delle cartelle. Vorrei chiedere al Governo come pensa che cittadini che non hanno pagato fin'ora con le rateizzazioni possano pagare ora dei debiti enormi in soli due anni; anzi, soltanto nel primo anno si deve pagare un importo pari al 70 per cento del debito complessivo. Il concetto è che, se facevano fatica a pagare prima, con una lunga rateizzazione, come faranno adesso? Andranno in banca a chiedere il prestito per pagare? E poi voglio vedere le banche che concedono il prestito. Inoltre rimane l'aggio per non dimenticare mai di remunerare Equitalia per il suo insostituibile servizio prestato alle casse dello Stato grazie grazie ai cittadini presi per la gola. Non è stata neanche prevista la possibilità di poter accedere a finanziamenti a tasso agevolato per debitori più in difficoltà. Vi ricordo che questi sono per lo più imprenditori che si sono ritrovati stretti nella morsa di Equitalia durante uno dei periodi più duri di crisi economica che questo Paese abbia mai attraversato. E tutt'ora

Ma cosa racconterà il Governo a quella parte di contribuenti che invece hanno già pagato, magari anche con innumerevoli sacrifici, stata per loro prevista, almeno, una forma di compensazione? Certo, questa misura non porta soldi immediati nelle casse di uno Stato come una manovra economica espansiva a *deficit*. E mi si potrebbe anche rispondere che le manovre espansive si fanno normalmente in *deficit*. Sì, è vero, ma non con la scure di una Europa evidentemente compiacente con un Governo che fa il suo gioco e che si può permettere di rinviare il pareggio di bilancio. nel caso, faremo in modo di avere forse un Governo migliore che aggiusterà i conti. Infine, vorrei fare un ultimo passaggio sulle disposizioni in materia di accoglienza. Come è possibile che il Governo si ostini nella sua assurda politica di accoglienza incondizionata per fare gli interessi di pochi che si arricchiscono con questo *business*? Più di 5.000 Comuni su 8.100 non aderiscono al sistema di accoglienza e il Governo è stato costretto a mettere delle mance nel provvedimento in esame pur di trovare una soluzione al ricollocamento dei migranti. E non solo offre un tot a migrante, ma consente anche a quei Comuni l'apertura di spazi finanziari. Sicuramente molti Comuni cederanno perché le politiche ai tagli operate da questo Governo li hanno prosciugati di moltissime risorse. Ma mi chiedo se non sarebbe stato più intelligente prevedere degli spazi finanziari per i Comuni in condizioni disagiate o interessati da situazioni di dissesto idrogeologico?

con i disegni di legge presentati da questo Governo. *In primis* c'è la finta abolizione di Equitalia.

io utilizzo proprio la parola «rubare», perché alcune sanzioni sono veramente esagerate. E allora disponete la rottamazione delle cartelle, ma non cambiate le norme successive e, quindi, create una disparità una disparità con chi ha pagato fin ad oggi. Non fate una distinzione tra loro che hanno veramente una difficoltà a pagare

Io no. Sono di oggi le parole di Alfano che difende il governatore De Luca sui toni usati e quello è un furbetto del quartiere. Vi stavo parlando della rottamazione delle cartelle. Bisognava fare un lavoro organico su Equitalia. Il rapporto del Fondo monetario internazionale e dell'OCSE deriva da un'interrogazione che evidenziava che i ruoli iscritti erano tantissimi: si parlava di 1.000 miliardi, quando in realtà quelli esigibili erano molti di meno, circa 50 miliardi. Allora c'è qualcosa che non funziona nel sistema, e non si può cambiare solo il nome, ma tutto il

È inutile che dite che rientreranno i capitali dall'estero e verranno pagate le sanzioni, perché è falso. un evasore riporta i soldi - mettiamo il caso li abbia portati nel 2003 o nel 2002 - per effetto della *voluntary*, l'Agenzia non potrà più verificare da dove derivano quelle entrate; potrà farlo solo sulla parte di maturazione di quei soldi.

e non quelle marchette che in ogni decreto-legge o in ogni legge di bilancio vengono inserite. Come non comprendere poi che questo decreto fiscale vi serve per il *referendum* costituzionale?

ne è la dimostrazione. Noi ormai abbiamo un Governo e una maggioranza che si ostinano ad andare avanti quando il popolo ha bisogno di altro. Il popolo italiano ha bisogno non di questo decreto, bensì di riforme organiche sul rapporto fisco-contribuente; non ha bisogno di una riforma costituzionale che non porterà alcun beneficio all'economia reale, come non aveva bisogno di quei decreti a favore delle banche. Vorrei ricordare il decreto Banca Italia e IMU,

fortemente contrario. Siamo veramente stanchi di lavorare in questo Parlamento, in questa Camera alta che viene utilizzata spesso dal Governo per i suoi incontri. È di qualche giorno fa l'incontro del

non dico consenzienti, ma certamente comprensive da parte dei rappresentanti della maggioranza. Questo decreto-legge avrebbe avuto ancora un mese di tempo per essere convertito in legge e viene convertito oggi: perché? Chi ha un minimo di esperienza parlamentare e di conoscenza dei modi di agire di questo Governo può immaginarlo. Abbiamo assistito negli ultimi anni all'immediato cambiamento di leggi appena approvate nelle leggi successive. Non è escluso che anche questo decreto, approvato domani in via definitiva con il voto di fiducia, possa essere oggetto di modifica

con una *dead line*, una linea di separazione, importante, che è quella del voto sul *referendum*. Un po' ironizzando, si potrebbe dire che siamo tornati ai tempi in cui, in alcune grandi città d'Italia, si facevano le campagne elettorali con le scarpe, dando la prima scarpa prima del voto e la seconda dopo il voto. Oggi il Governo ci fa ricordare quei tempi: prima del voto dà un decreto-legge e mezza legge di stabilità;

il secondo era l'abolizione di Equitalia; il terzo era una riapertura dei tempi del volontario rientro dei capitali, con le conseguenze penali, che portano soldi nelle casse dello Stato. Sono stati affrontati questi tre argomenti dal Governo, ma in che modo? In modo assolutamente sciatto - mi sia consentito - perché l'abolizione di Equitalia è solo una norma manifesto.

d'esecuzione, che privilegiano gli incassi da parte di Equitalia sulle ipoteche, sulle procedure forzate, su tutto quello che è strumento di vessazione nei confronti dei cittadini. Invece, si si rottamano le cartelle, nel senso che si può pagare la sola sorte capitale, ma si mantengono le condizioni affinché da qui a qualche anno il monte di impagato, dovuto all'eccesso delle sanzioni, degli interessi e degli aggi, si ripresenti e si debba fare lo stesso provvedimento; e si ripresenti con tutte le negatività che in corso d'opera si registrano circa il disagio dei contribuenti e la loro assoluta preoccupazione, in un Paese che continua ad avere la più alta pressione fiscale. Peccato che il Presidente del Consiglio se ne sia accorto solo questa mattina: ha fatto una dichiarazione alla scuola della Guardia di finanza dicendo che è intollerabile che il nostro Paese ha la più alta pressione fiscale d'Europa. Ma lui è in campagna elettorale, come qualcuno che non ha mai messo piede in Parlamento - questo è vero - o è Presidente del Consiglio da tre anni? E questa considerazione non se l'è mai posta?

addirittura configurano degli scambi elettorali con pezzi del proprio stesso partito (vedi il caso Campania) o con fasce di popolazione, perché poi questo Governo non è neanche capace di fare le cose buone che vorrebbe magari fare (diamogli il beneficio della buona volontà). Organizza una semplificazione burocratica che è, invece, una complicazione, tant'è che tutti gli ordini professionali

Sono sul piede di guerra gli spedizionieri doganali, che si sono visti cambiare le norme sull'Intrastat e denunciano che nel cambiamento di norme si annida una clamorosa evasione fiscale dell'IVA infracomunitaria. Non so se si tratta di cattiva volontà o del fatto di essere maldestri. Certo è che tutti questi provvedimenti continuano a suscitare la reazione degli addetti ai lavori. dei provvedimenti spiccioli. Il Governo e la maggioranza, soprattutto la grande maggioranza della sinistra che ha i suoi principi inattaccabili, ci hanno sempre detto che non avrebbero mai fatto condoni. parte il fatto che questo è un condono: anche se non incide sul *quantum* del capitale, certamente crea una profonda disparità tra chi ha pagato anche con un minimo di interessi e chi domani pagherà senza neanche un centesimo di interessi. Ma lasciamo perdere, e su questo noi potremmo anche convenire. Tuttavia l'articolo 5-*bis*, introdotto alla Camera, consente un condono solo alle grandi società I colleghi sanno bene quali sono i rapporti tra il Governo e le società petrolifere. Sanno bene che basta scorrere - ove mai dovessero essere pubblici - gli elenchi dei partecipanti alle cene di finanziamento del Partito Democratico per sapere chi sono i facoltosi depositari dei 30.000 euro a posto per potervi partecipare. Guarda caso: spunta un clamoroso condono (nel senso tecnico della parola) per le grandi società petrolifere, che possono

di quei cittadini che non hanno pagato per motivi di necessità, per motivi dovuti al loro stato economico personale? casi non si trattava di un'evasione, ma di un non pagamento per stato di necessità. Certo, qualcuno utilizzerà sicuramente la rottamazione, perché una cosa è trovare i soldi per pagare 40 e una cosa è trovarli per pagare 10; questa è normalmente la differenza, sulle cartelle esattoriali, tra il capitale e tutto il cumulo delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.

(cartelle, rientro dei capitali e abolizione di Equitalia). Ma tutto è stato stravolto; ancora una volta tutto è stato condizionato e piegato alle strategie ormai machiavelliche del Governo per cercare di ottenere un minimo di consenso al *referendum*. Ma, io, invece penso che gli italiani sapranno con molta saggezza rifiutare una proposta

evasione fiscale, di essere equo nei confronti del cittadino e di produrre effetti positivi per la finanza pubblica, le modifiche sono state sempre molto poche e sempre molto misurate e solo oggi abbiamo una corposa riscrittura di questa tematica. Ovviamente sto

Il risultato di questa vicenda è noto, è pubblicato sistematicamente, viene richiamato in modo puntuale da tutti gli organi che si occupano di finanza pubblica e di gestione dell'economia

la certezza del condono fiscale. Questi tre elementi costituiscono la ragione stessa per la quale abbiamo la dimensione dell'evasione fiscale

introduce una sorta di norma programmatica strana, in cui si dice che Equitalia non esiste più, ma l'ente strumentale che la dovrà sostituire nell'attività di riscossione esisterà tra circa sette mesi, dal primo di luglio. Nel frattempo organizza questo trasferimento di competenze che appare uno dei tanti traslochi che siamo capacissimi di promuovere per creare confusione. Signor Presidente, non so se lei ha mai cambiato casa, se ha mai gestito un trasloco, se ha mai riempito le scatole, poi svuotato le scatole o lasciato le scatole piene senza mai svuotarle nel tempo, pur avendo cambiato casa. che devono essere invece puntualmente esercitate, perché, guarda caso, quello è l'ente che deve provvedere alla provvista finanziaria per reggere il bilancio dello Stato. Noi facciamo un trasloco

in un momento in cui - badate bene - la condizione economica e la salute delle casse dello Stato non è tra le migliori, ma, anzi, è una situazione di evidente crisi e difficoltà. Non possiamo quindi introdurre in questa fase un elemento aggiuntivo di difficoltà. Non so cosa succederà, ma lo posso immaginare: succederà esattamente quello che è sempre successo quando abbiamo promosso questi processi. L'unica cosa che funzionerà, Presidente, è il sistema di condoni rispetto all'obbligo di pagare le imposte che qualcuno non ha osservato. La seconda cosa che succederà, signor Presidente, è che chi ha pagato, chi ha svolto in modo pieno la propria funzione di cittadino contribuente, ovviamente sarà invogliato ad aspettare il prossimo trasloco per godere dei benefici di un ulteriore condono rispetto all'adempimento degli obblighi fiscali.

fiscale. Dobbiamo avere le idee chiare su qual è questa funzione e come va esercitata. Dobbiamo dare non l'incertezza del diritto che abbiamo dato fino a oggi e che ha avvantaggiato i privilegi e i privilegiati, ma dobbiamo finalmente tutelare i grandi contribuenti, che - badate bene - sono i piccoli sono i lavoratori dipendenti, quelli che hanno la busta paga sotto controllo, quelli che fanno il proprio dovere di lavoratori autonomi, rispondendo in modo sistematico alle leggi che regolano il contributo alle casse dello Stato. Stiamo parlando degli onesti: gli onesti sono puntualmente turlupinati da questo modo di comportarsi del Parlamento e dei governi. Non va bene più più lo abbiamo detto e lo ripetiamo: gli unici che godono sono i privilegiati che fino a oggi hanno avuto privilegi. Dobbiamo pensare che la certezza del diritto, sopratutto in materia fiscale, è la ragione stessa della condizione di rispetto del cittadino e dei suoi diritti, nel quadro dei suoi doveri. Violare questo principio vuol dire violare la Costituzione, cioè il dovere-diritto del cittadino a contribuire allo sviluppo della propria comunità nazionale, così come è sancito nella parte fondamentale della

Presidente, colleghi senatori, siamo chiamati al sessantaquattresimo voto di fiducia in poco più di mille giorni, un vero *record* negativo di questo Governo. in esame è in pieno contrasto con l'articolo 77 della Costituzione, che prevede per tale strumento gli indispensabili requisiti di straordinarietà, di necessità e di urgenza, requisiti che non si ascrivono a questo provvedimento. il voto di fiducia su cosa è? Di certo non sulla tanto proclamata rivoluzione del sistema fiscale e di riscossione delle imposte. Purtroppo, è solo l'ennesima prova dell'arroganza di Palazzo Chigi, che calpesta ripetutamente le prerogative del Parlamento per accentrare anche il potere legislativo nelle mani del Presidente del Consiglio. Un *one man show* che fa propaganda elettorale h24 presentando *spot* i cui contenuti sono, però, sempre molto diversi dagli atti sottoposti alle Camere per la sola presa di conoscenza. Oltre alla forma, è nel contenuto che si manifestano le più grandi contraddizioni, a cominciare dalla soppressione di Equitalia. Questa è solo l'ultima presa in giro degli italiani, come già fatto con i proclami su Province e Senato. La soppressione cela solo una sua mera trasformazione da società a partecipazione pubblica ad ente pubblico economico, che fa capo alla Presidenza del Consiglio. Ecco, quindi, qual è l'obiettivo vero: conferire al *Premier* il potere di controllare anche questo comparto. Una vera riforma di riscossione delle imposte era stata varata dal Governo Berlusconi nel 2005 ma la sinistra, con il presidente Prodi, ha stravolto quanto di buono era stato fatto, creando quel mostro di Equitalia che tanti danni ha fatto agli italiani. Non è cambiando il nome che si risolvono i problemi dei nostri concittadini. Addirittura, oggi questa nuova Agenzia ha poteri molto più pervasivi che le permettono l'accesso alle banche dati dell'INPS. Anche sulla rottamazione delle cartelle esattoriali abbiamo ascoltato solo menzogne. In realtà, è prevista solo la possibilità di dilazionare il pagamento in un massimo di cinque rate entro il 2018. Questo provvedimento è pensato esclusivamente per fare cassa a tutto vantaggio degli evasori e, come sempre, a scapito dei contribuenti onesti ma in difficoltà. Forza Italia, al contrario, ha presentato un disegno di legge che prevede uno scaglionamento dei debiti tributari attraverso un piano di rientro. La proposta tiene conto degli interessi degli italiani, pur riuscendo a soddisfare anche gli interessi di bilancio. Inoltre, anziché semplificare, si aggiungono ulteriori adempimenti in capo alle aziende, come la dichiarazione trimestrale di tutte le fatture ricevute ed emesse, come se non fossero sufficienti le 269 ore spese di media dalle nostre imprese per adempiere agli obblighi burocratici, con un costo per le stesse imprese pari a 30 miliardi che porta il nostro Paese al 44o posto nel *ranking* annuale sulla competitività stilata dal World Economic Forum. Infine, dopo aver fatto cassa sulle spalle degli italiani è negli articoli finali che Palazzo Chigi dà il meglio di se stesso prevedendo una serie di elargizioni a pioggia ai soliti amici degli amici: dal finanziamento a Ferrovie dello Stato per investimenti ai trasporti campani e molisani, alle norme che concedono fondi ai Comuni alle prese con l'accoglienza dei migranti, infine al *tax credit* per il cinema. Il decreto-legge in esame ha la stessa natura delle sirene affrontate da Ulisse nel poema «Odissea». Infatti, proprio come quelle creature mitologiche che blandivano i marinai per poi attaccarli senza pietà, con questo provvedimento il Governo tenta di blandire gli italiani con un titolo ad effetto, al fine di occultare le mostruosità, se non addirittura le pericolosità, contenute al suo interno. Ma gli italiani oramai sono immuni alla retorica renziana e ne daranno prova il prossimo 4 dicembre.

velocemente e aiuta la regolarizzazione delle insolvenze. Vi è però un primo problema, perché quanti sono effettivamente gli evasori, dolosi o colposi, e i distratti e quanti invece gli incapienti che non possono pagare? Oggi Equitalia permette la rateizzazione delle cartelle esattoriali in 72 rate mensili, ossia sei anni.

i ravveduti in buone condizioni, ma non per chi è in crisi vera. Infatti, chi versa in crisi vera e non riusciva a rispettare il termine dei sei anni, di sicuro non riesce a saldare il debito in un anno e mezzo. È fin troppo semplice.

adempimenti all'anno (spesometro trimestrale e comunicazione dell'IVA trimestrale). Alla faccia della semplificazione! Alla faccia del bicarbonato di sodio, che ci sarebbe da prendere! Allora, per curiosità, ho contattato alcuni commercialisti e ho chiesto quanto

l'Agenzia delle entrate fa fare lavoro pubblico a dei privati, con un costo, perché questo ha un costo che ricade sulle imprese e sulle partite IVA; e se non ricade sulle imprese e sulle partite IVA vuol dire che i commercialisti dovranno lavorare

aggravio farà sparire le imprese; i clienti non possono pagare di più, quindi spariscono proprio. Questo è un modo per distruggere il lavoro autonomo, la piccola impresa, cioè tutto quello che fa lavoro concreto, la buona Italia, quella veramente buona: quella che non lavora sulla burocrazia quella che non si ritrova senza meriti nel pubblico, senza concorso, con uno stipendio «strapieno». Quella che, al contrario, è abituata a conquistarsi le cose giorno per giorno, si trova ulteriormente

acquistato un *software* privato che avrà un costo. Mi ricorda tanto quello che è successo per i medici competenti, per l'allegato 3B: i dati di rilevamento epidemiologico in capo alle ASL vengono estrapolati e affidati a medici liberi professionisti che fanno il lavoro gratis. Questo è un modo per dare al pubblico del lavoro gratuito fatto da privati. Dico, allora, una cosa molto semplice: l'estrapolazione dei dati dalla contabilità deve essere automatica e

tutte le fatture di acquisto e vendita passive e attive. Questo processo mi ha ricordato la rendicontazione assurda del «tirendiconto» dei 5 Stelle, in cui uno doveva presentare tutti gli scontrini;

allora, non si può alzare*, random*, e fare i controlli che ritiene sulla base di altri criteri? Da quando in qua fare attività fisica, alzarsi dalla sedia e muoversi è una controindicazione per la salute?

Io volevo restasse agli atti che questa non è semplificazione, quella che noi chiediamo e che io chiedo da sempre. La semplificazione vera va fatta diversamente e non deve essere a carico dei privati. *(M5S)*. Signor Presidente, questo decreto fiscale mette insieme capre e cavoli, come sempre sotto l'egida della somma urgenza o, se preferite, della solita fretta che, come sempre, porta solo danni al Paese e favorisce, in maniera nemmeno troppo velata, il clientelismo e forse anche il voto di scambio. Come non notare, signor Presidente, che all'interno dello stesso provvedimento, si riscontrano materie troppo differenti tra loro per essere messe insieme e che di urgente non hanno proprio nulla, se non la fretta del *Premier* di distribuire mancette per accaparrarsi qualche voto in più al *referendum*, a partire dalle false speranze alimentate dall'annunciata chiusura di Equitalia, che in realtà cambia solo nome, e potenzia invece gli strumenti di accertamento e riscossione, con buona pace delle piccole e medie imprese? Cosa c'entra, poi, la missione Ippocrate con il fisco? L'articolo 9, infatti, stabilisce misure per il finanziamento di questa nuova genialata in Libia, che fa dell'Italia l'unico paese a stanziare truppe regolari nel Paese, a difesa di un ospedale militare creato per curare i miliziani di Misurata, pesantemente sospettati di alimentare il traffico di esseri umani dalla Libia e non solo. È bene ricordare ai presenti e ai cittadini a casa, che questa storia dell'ospedale di Misurata è divenuta nel frattempo obsoleta: Al Sarraj non detiene il potere che in Italia i nostri Ministri degli esteri e della difesa dicono abbia. La situazione in Libia è cambiata velocemente, minando ulteriormente il "prestigio" di questo eterno "*premier* designato" ed esponendoci a ritorsioni che prima o poi metteranno alla prova i nostri uomini in Libia. Va ricordato che le milizie di Zintan, tra le più potenti nel Paese, a fine ottobre ci hanno già chiamato invasori neo coloniali e che presto o tardi catalizzeranno altri gruppi per farci la guerra. Perché spendere 17 milioni solo per il 2016 per rischiare ritorsioni? Sarà certamente al corrente il nostro Ministro degli esteri che la stessa Tripoli non è sotto il controllo di Al Sarraj e che la situazione volge a favore del Parlamento di Tobruk e di Haftar che, una volta conquistati i terminali petroliferi di Ras Lanouf, ha ipotecato il controllo della Libia, almeno per il momento, a scapito del traballante Al Sarraj. Sottolineo sommessamente che la campagna elettorale americana è finita che non è più necessario dimostrare al mondo che gli USA di Clinton e Obama e gli alleati vogliono combattere un surrogato dell'ISIS, visto che in altri posti, ad esempio ad Aleppo, si sostengono soggetti uguali se non peggiori a quelli che si stanno combattendo in Libia, con buona pace della coerenza. Ancor più contraddittorio è il fatto che noi sosteniamo un'altra milizia islamica, quella di Misurata, che in quanto a pratiche efferate, non ha nulla da invidiare ai più famosi cugini dell'ISIS, che pure combatte a Sirte. Certo, dovremmo ammettere che abbiamo puntato sul cavallo sbagliato, ma è forse conveniente perseverare nella costruzione di un ospedale militare, senza nemmeno prevedere sistemi di sostegno medico alla popolazione libica, stremata da anni di caos di cui anche l'Italia è responsabile? Dobbiamo necessariamente mettere in pericolo le nostre forze in una missione in cui, lo ripeto ancora una volta, gli unici ad aver schierato truppe regolari siamo noi? Noi siamo sicuramente disponibili ad ascoltare in Aula le strategie del Ministro degli esteri - lo facciamo con Renzi, figuriamoci - però francamente finanziarle pure, mettendo a rischio la vita dei nostri valorosi militari e dei medici è davvero troppo. Vi facciamo una proposta: questi 17 milioni utilizzateli per la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica e in cambio a Natale vi regaliamo un bel Risiko, così potete giocare alla guerra senza fare danni all'Italia e alla Libia. Andiamo avanti: l'articolo 10 finanzia gli investimenti per le Ferrovie dello Stato. Domanda: era questo decreto-legge detto fiscale, quello giusto a finanziare un'esigenza sicuramente avvertita, ma non imprevedibile? L'articolo 11 reca misure urgenti per il trasporto regionale, che non riguardano tutte le regioni, ma solo la Campania con 600 milioni e il Molise con 90 milioni. È da sottolineare che c'è una stretta relazione tra il De Luca della riunione del 15 novembre con i trecento sindaci, in cui illustra una pioggia di milioni da parte del Governo e a cui rispondere con un voto di massa per il sì al *referendum*, e l'improrogabile necessità che stiamo discutendo oggi. Noi, francamente, vediamo solo la necessità di raccattare voti al *referendum*, fidelizzando definitivamente "chi il clientelismo lo sa fare come Cristo comanda": e non sono parole mie. Eccoci dunque al plateale smascheramento del voto di scambio: il Governo appiana seicento milioni di debiti e De Luca mobilita i sindaci per procurare voti per il *referendum*: all'ultimo articolo, il 15, signor Presidente, anche in questo caso è singolare che un decreto fiscale, discusso in fretta e furia, si occupi di questi temi. Allora perché lo avete chiamato decreto fiscale? Potevate chiamarlo legge di stabilità, almeno sarebbe stato più coerente.

questo decreto-legge merita l'appoggio del Gruppo Partito Democratico e quindi la fiducia al Governo che lo ha proposto. In un Paese dove, come abbiamo avuto conferma anche oggi pomeriggio, il "benaltrismo" è il *leit motif* prevalente per contrastare ogni tipo di decisione, questo decreto-legge è un provvedimento concreto, sia per lo Stato che per il cittadino. Contribuisce in modo significativo alla manovra di finanza pubblica 2017-2019, cui è collegato, prevede maggiori entrate, considerata anche la riproposizione della *voluntary disclosure,* per circa 16 miliardi di euro nel triennio. Queste maggiori entrate sono il frutto dell'attivazione di nuove azioni, volte a migliorare il rapporto tra fisco e contribuente, attraverso un nuovo ruolo attribuito all'amministrazione fiscale. Modulare in modo più flessibile il comportamento del fisco a seconda che si tratti di errori "colposi" dei contribuenti o di suoi intenti "dolosi" o "fraudolenti"; gli strumenti della comunicazione moderna (SMS e PEC) per segnalare criticità ai contribuenti e invitar loro a spiegare situazioni poco chiare; promuovere, cioè, una *tax compliance* dei contribuenti al posto del burocratico e vessatorio approccio che tutti abbiamo conosciuto, è un passo in avanti per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nella delega fiscale e che troveranno ulteriore conferma e disciplina nella riforma del processo tributario e nel più diffuso utilizzo degli strumenti elettronici. È in questo contesto che si inquadrano anche la soppressione di Equitalia, la cosiddetta "rottamazione delle cartelle", le norme su una maggiore semplificazione, l'introduzione della comunicazione trimestrale, finalizzata a superare il "*tax gap* IVA" (il rapporto cioè tra tassazione potenziale ed effettiva che nel nostro Paese è molto ridotta rispetto al resto d'Europa) che è compensata dalla soppressione dell'obbligo di comunicazione dell'elenco fornitori e clienti, il cosiddetto spesometro, ed altri minori adempimenti, che rendono del tutto ingiustificabili e immotivate le critiche, anche del mondo delle professioni, nei confronti

telematici, quando invece, forse, con un *click* è più facile risolvere i problemi che facendo polemiche. Si dà in sintesi attuazione a quella strategia "cambia verso" annunciata dal Governo, che non elimina la riscossione ovviamente. Ma dove non esiste la riscossione? Si dice che non elimina le sanzioni. Ma dove non esistono le sanzioni per chi evade e per chi elude? Ma il provvedimento riconduce tutto a quell'essenziale e fondamentale contratto sociale che lega il cittadino allo Stato. Uno Stato che punisce chi evade e chi elude, ma che agisce con prudenza, disponibilità e tolleranza verso chi sbaglia senza dolo o che si trova in momentanee difficoltà economiche ma è in grado di assolvere ai suoi impegni, magari chiedendo dilazioni. In parte, norme di questo genere dal punto di vista del loro presupposto culturale appartengono già alla nostra normativa. Il problema è andare progressivamente verso una maggiore semplificazione e un approccio migliore tra cittadino e contribuente. Non condoni, quindi, ma interventi volti a ricostruire un rapporto fiduciario, da tempo compromesso e che va ripreso nell'interesse di una maggiore coesione sociale. sociale. Senza entrare nel dettaglio di ulteriori aspetti, anche citati oggi, di questo decreto fiscale, questi sono i motivi e le ragioni di fondo che lo rendono urgente, non nel senso letterale del termine, anche voluto dalla Costituzione, ma urgente rispetto alle dinamiche del nostro contesto sociale; in ogni caso rispettoso del dettato costituzionale, ma non limitiamoci agli aspetti formali. C'è una urgenza maggiore, che è quella che ci giustifica nel dire sì a questo provvedimento. Signor Presidente, vorrei approfittare del tempo prezioso dei colleghi,

le valutazioni che vedo che già in questa sede vengono svolte da alcuni colleghi sul piano più politico.

quello che, soprattutto nell'attività e nell'azione di questo Governo, porta a nascondere sotto mentite spoglie nuovi strumenti di pressione fiscale. Si tratta in effetti

complessivamente, tra la lettura della Camera e quella del Senato, credo abbia tenuto impegnato il Parlamento per trentuno giorni. È un provvedimento che individua nel proprio cuore il valore di quel fisco amico che in molti rincorriamo? Direi di no. Altro che *tax compliance*, collega Susta. Non lo è per nessuno, ma in particolare

C'è invece per le partite IVA, per i professionisti, ma anche per tutti i contribuenti un aggravio di procedure che la senatrice Fucksia prima ha persino descritto nel loro valore economico, indicando cioè quanto costerà a questi soggetti farsi carico di ulteriori spese di ulteriori spese e oneri per poter restare almeno in contatto con il fisco. Altro che fisco amico! ancora una volta alla propaganda; una propaganda che, tanto per rimanere alla parte del testo su Equitalia, che enfaticamente viene annunciata come abolita, è invece funzionale e rendere più stringente il rapporto tra fisco e cittadini. Prima ancora della *tax compliance* io vorrei semplicemente vedere rispettato quel codice

nasconde al proprio interno un comodo condono e consiste in una finta dilazione, che converrà solo a chi a chi ha già i soldi per poter regolarizzare la propria posizione con il fisco attraverso Equitalia. Infatti, chi non aveva quei soldi, non certo per colpa sua ma a causa di una crisi gravissima che si è abbattuta sulle nostre piccole imprese, sui lavoratori autonomi e sulle famiglie, ieri poteva godere di una dilazione nel pagamento, di una rateizzazione nei pagamenti verso Equitalia che arrivava a oltre sei anni,

Quindi noi non siamo alle prese con un buon decreto fiscale: noi siamo alle prese con un decreto-legge *omnibus*, che utilizza la scusa del decreto fiscale per fare altre cose, ma soprattutto per per portare non solo ulteriori aggravi ma ulteriori dolori a quei contribuenti che avranno di che accorgersi molto presto di ciò che si nasconde dentro questo decreto fiscale. Ad esempio, quel testo che dovrebbe impedire l'uso dei dati dei contribuenti per fini diversi da quelli statutari non è scritto, mentre invece avremmo dovuto avere molto a cuore quello che determinerà l'utilizzo delle banche dati e l'incrocio di tutti i dati e delle informazioni in questo grande moloch che oggi diventa l'assorbimento da parte dell'Agenzia delle entrate anche dell'ente della riscossione Equitalia. Equitalia. Ulteriori aspetti più controversi riguardano: il recupero delle accise in caso di fallimento, perché riusciamo a far pagare le tasse anche ad aziende che sono già fallite. della platea dei soggetti che possono avvalersi della rottamazione delle cartelle, prevedendo ad esempio un massimo di dodici rate trimestrali per effettuare il pagamento (era una delle proposte che da parte di più Gruppi saliva); che la rottamazione delle cartelle non sia valida se il pagamento avviene per tre rate anche non consecutive (oggi invece è limitata a una sola rata); il fatto che il mancato pagamento di una rata non produce la decadenza se il debitore dimostra difficoltà economica; il fatto che gli effetti interruttivi del mancato pagamento decorrono dalla data di presentazione della domanda relativa ai ruoli o alle cartelle.

persino la voce dei pignoramenti ai cittadini e contribuenti italiani nel valore stimato dalla Ragioneria generale dello Stato in 500 milioni. Noi utilizziamo 600 milioni per alcune delle iniziative che hanno il vago sapore elettorale in questa fase da parte del Governo, dandogli la copertura dei pignoramenti che verranno fatti agli italiani che fino ad oggi hanno potuto contare su una rateizzazione e che da domani non potranno più Concludo il mio intervento ricordando come quel tema ossessivo del controllo persino del prelievo del proprio denaro - lo ha detto bene prima di me e meglio di me il senatore Tremonti ci metta di fronte a una grande riflessione. Nei giorni della crisi bancaria più drammatica della storia del nostro Paese, noi non siamo affatto preoccupati da quel dettato costituzionale che ci impone la tutela del risparmio, valore costituzionalmente garantito nel nostro Paese. Come apprendiamo dal decreto fiscale del Governo, siamo invece molto, molto preoccupati dalla disciplina del risparmio e di come dobbiamo costringere gli italiani ad utilizzare il loro denaro; se possono o se o se non possono prelevarlo; se possono utilizzarlo nella libertà della loro proprietà oppure no. Ecco, questa è la vostra Costituzione alla rovescia: la tutela del risparmio no, ma il controllo del risparmio sì. Questo ci porta a definire questo decreto fiscale l'ennesima occasione perduta per poter davvero andare verso quel fisco amico che forse in questo Paese non vedremo mai. Signor Presidente, siamo all'ennesima fiducia da parte del Governo. Credo correrebbe l'obbligo di farci la compiacenza di numerarle, di volta in volta, per avere un quadro generale del numero. Signor Presidente, che la questione fiscale abbia un ruolo centrale nella vita economica di tutti i Paesi avanzati, e in particolare in Italia, è cosa nota a tutti. Il Governo, con il decreto-legge che stiamo esaminando, cerca di mettere ordine sull'intero comparto. Ciò, purtroppo, non avviene nella direzione che sarebbe auspicabile, vale a dire abbassando decisamente le imposte sulle attività produttive e sui redditi da lavoro e colpendo invece con decisione le rendite e le ampie sacche di evasione ed elusione; avviene attraverso una serie di provvedimenti demagogici e dal sapore elettoralistico: spicca fra tutti, la vantata abolizione di Equitalia. In vista del *referendum* si vuol far credere che verrà abbattuto il mostro odiato da intere categorie, l'ente che è stato presentato come la causa di tutte le disgrazie nazionali. In realtà, secondo un costume abituale nel Paese delle grida manzoniane, ci si appresta a cambiare non la cosa, ma soltanto il suo nome. Non Equitalia, ma le targhe dei palazzi dove Equitalia ha sede. Il nuovo ente sarà tenuto a conformarsi alle stesse regole di prima, dovrà applicare le stesse percentuali negli oneri di riscossione e negli interessi di Inalterata, naturalmente, resterà la dirigenza. Gli unici a essere penalizzati dal cambiamento saranno, probabilmente, i dipendenti, additati come capri espiatori per aver applicato regole non da loro stabilite. Altrettanto negativo appare la norma sulla cosiddetta *voluntary disclosure*, grazie a cui, con il pagamento di una piccola tassa, coloro i quali detengono denaro contante all'estero potranno riportarlo in Patria. Dietro la cortina fumogena, ormai diventata abituale, di una altisonante espressione inglese si nasconde l'ennesima squallida sanatoria. Ancora una volta, lo Stato italiano si accinge a condonare, con una pacca sulla spalla, chi ha accumulato fortune evadendo il fisco, o, ancora peggio, dedicandosi ad attività criminali: pensate un po', sarà lo Stato stesso a lavare i soldi sporchi! Tutto questo mentre invece i giovani artigiani o coloro che cercano di avviare una piccola impresa non avranno alcuna agevolazione. Per fare un esempio, i costi dell'avvio di una nuova attività per chi possiede capitali limitati o non ne possiede a sufficienza sono sempre troppo onerosi e possono arrivare, nella migliore delle ipotesi, fino a 15.000-20.000 euro. Ricordo infine la norma con cui vengono stanziati 600 milioni di euro per l'accoglienza dei profughi. Si tratta di un classico intervento palliativo, in un momento in cui i centri di accoglienza sono sovraffollati, i migranti si trovano a vivere in condizioni di degrado destinate a favorirne, nel medio periodo, l'arruolamento nelle associazioni criminali e mentre la loro ricollocazione in luoghi più idonei (in Italia, all'estero e soprattutto nei Paesi di provenienza) neppure è tenuta in considerazione. Insomma, si stanziano soldi senza la predisposizione di regole, che invece sarebbero assolutamente necessarie. Potrei fare altri esempi, ma sarebbe superfluo. Il nocciolo della questione mi sembra già abbastanza chiaro: questo decreto-legge aiuterà forse il Presidente del Consiglio a raccogliere qualche migliaio di voti in più nel *referendum* del 4 dicembre, di sicuro non aiuterà l'Italia ad uscire dalla sua drammatica crisi.

Signor Presidente, sarò molto breve, anche se sono cosciente che - con tutto il rispetto per i colleghi presenti - parlo a un'Assemblea che è diventata sorda, assente e, nella gran parte dei casi, assuefatta. Siamo qui a discutere di un decreto fiscale che ha un unico obiettivo: fare cassa

penso che, se il Governo fa questi interventi sotto l'aspetto elettoralistico, di politica elettorale comprende molto poco, soprattutto perché ha irretito tantissimi cittadini italiani che, come me, aspettavano con ansia questo decreto-legge;

menzione, signor Presidente, di quello che già tanti colleghi hanno detto prima di me: di Equitalia, di quello che si farà di Equitalia e di tutto quanto è accessorio, anche se di grande sostanza.

Perché dico questo? Perché al comma 1 dell'articolo 3 si dice: «A decorrere dal 1º gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla

avrebbe carpito probabilmente la buona fede di tanti cittadini; invece, stupidamente, lo converte oggi, facendo comprendere loro che non potranno risolvere i loro problemi di natura economica e di ripristino delle posizioni personali rispetto al fisco. Bandirei, quindi, questo aspetto strumentale ed elettorale,

noi ci ritroviamo con un provvedimento nel quale alla Camera è stato inserito l'articolo 5-*bis*, con il quale ai petrolieri, ai produttori di tabacco e ai produttori di alcool si concede

grave. Infatti, alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 5-*bis*, si dice che «al soggetto passivo d'imposta è data facoltà di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20

mio Gruppo politico - il riferimento al sindaco di Eboli, per quanto riguarda le fritture, probabilmente deriva da un *lapsus* freudiano,

per le diverse cose che ho detto poc'anzi e per le tante altre che potrebbero ancora dire, ma, ahimè, il tempo è tiranno e mi devo rifare alla dichiarazione di voto del mio Capogruppo nella

La seconda storia di ordinaria follia che voglio raccontare in quest'Aula è la politica economica che sta portando avanti il Governo e la modalità con cui la sta portando avanti.

Tra l'altro, sempre in base alla modifica che avete approvato, la legge di contabilità non permetterà più il controllo dei flussi di denaro: e questo è un grosso problema, che già aveva evidenziato la Corte dei conti. Quindi, questo è un decreto-legge che non solo funge da copertura alla legge di bilancio, è anche un collegato alla legge di bilancio, ma è un provvedimento che non rispetta assolutamente la legge di contabilità, per svariati motivi. Il primo motivo

era inserito nelle tabelle della legge di bilancio, vuol dire che queste coperture *una tantum* serviranno per coprire le spese della legge di bilancio. Peccato che prevediate coperture *una tantum*,

pura. In secondo luogo, queste coperture non sono quantificate, sono soltanto una previsione: altra follia. Infatti, una copertura per la legge di bilancio deve essere non solo quantificata, ma anche correttamente quantificata, altrimenti la legge di bilancio non sta in piedi. Il terzo motivo per cui non rispetta la legge di contabilità è la questione delle quote che derivano dalla lotta all'evasione fiscale: i soldi che arrivano dalla lotta all'evasione fiscale devono essere collocati nel Fondo per l'abbattimento della pressione fiscale. Mi rivolgo al Governo: non è che basta inserire la parola «fiscale» nel decreto-legge

Vorrei spendere poi due parole sulla lotta all'evasione fiscale. Mi sono un po' stancata di sentire che lottate contro l'evasione fiscale solo a fine anno,

per cento. Se fosse fatta una lotta seria alla corruzione, avremmo i lavori pubblici che costerebbero meno e lo Stato avrebbe soldi in più da investire per gli italiani. Inoltre, i principali investitori esteri

avete sterilizzato 15 miliardi di clausole di salvaguarda. Questi non sono gli ultimi miliardi di clausole di salvaguardia, che vengono

la penosità fiscale di quelle cartelle assoggettate a sanzioni irragionevolmente onerose. Quindi, è un provvedimento che bene ha fatto il Governo adottare questo provvedimento sarebbe stato necessario fare soltanto una cosa: modificare la norma che dà luogo a quelle sanzioni onerose e che gonfia quella che definirei, impropriamente, la sovrattassa di riscossione. riscossione. Si poteva vessare meno i cittadini e trasparentemente cogliere l'occasione per il pregresso.

No. L'ottimo Governo Renzi, pur di guadagnare un po' di pubblicità (non di più, perché, come vedremo, le malefatte in tanti ambiti sono parecchie e alcune verranno presto

trasporta il personale, mantenendo situazioni che già ci sono e, portandole non si sa come, le riattribuisce all'Agenzia delle entrate-Riscossioni, che però riscuoterà direttamente, ma attraverso un nuovo ente strumentale che non so come si chiamerà. L'ente strumentale per definizione subentra a titolo universale in tutti i rapporti giuridici e riecco

«Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.» ossia tutto quel che ho appena

e da domani continuate come prima. Ma non vi preoccupate, ho cambiato il nome! E poi fa un pasticcio, capirete, con passaggi di personale e quant'altro, che naturalmente troveranno tutta una serie di problematiche che al momento non siamo in grado di vedere, ma che certamente sorgeranno. Una cosa che, davvero, nemmeno nemmeno la peggior fervida immaginazione poteva pensare! Quindi, diciamo agli italiani che gli facciamo una cosa solo per il passato e

ora davvero può essere buona questa norma? No! E prevede solo quattro rate, poi diventate cinque con il passaggio alla Camera, per cui, un signore che aveva spalmato il suo debito in sei anni lo deve pagare in un anno, seppur con una riduzione del 30 per cento. È vero che sarà possibile accedere a forme di finanziamento, ma questo fa parte della saggezza, dell'astuzia del cittadino che si ingegna e trova la strada. Il Governo non ha tenuto in piedi nemmeno l'unica cosa buona che avrebbe potuto tenere. E attenzione: poi, le cinque rate diventano un vezzo, e il Parlamento, che dopo il 4 dicembre non sarà chiuso ma sarà ancora aperto, provvederà a fare qualcosa in favore dei cittadini. Questo è davvero ciò che è accaduto, testo alla mano.

dialetto, credo *talk show* (o una cosa del genere). Ebbene, nei *talk show* non si dice niente di tutto questo e si inventano cose terribili e si specula sul terribile dramma di chi si vede sanzioni straordinarie e l'unica cosa che vuole è che si abolisca il nome Equitalia, ma noi abbiamo il dovere di essere lucidi e fare davvero gli interessi del cittadino.

Prego tutti i senatori e le senatrici di vedere la pagina della relazione tecnica che correda questo provvedimento e che illustra gli adempimenti a cui saranno soggetti i cittadini in base a questo decine e decine; riempiono tre pagine e si intersecano in maniera incredibile. Naturalmente sono già insorti tutti (se ne stanno accorgendo: attenzione, è pericoloso!) perché naturalmente diverrà un costo in più per chi paga le tasse, perché sia che l'impresa grande debba potenziare i suoi uffici addetti per dar corso a questi adempimenti, sia che le imprese più piccole ricorrano a consulenti, sono costrette a dover pagare di più.

Per di più, da questo viavai di carte - immaginate quante, dirò qualcosa in proposito - si prendono centinaia di milioni in più: che gioia per questi cittadini che pagano ulteriori centinaia di milioni di tasse! Siete fantastici! Dite ai cittadini che con questi nuovi adempimenti ritenete di adempimenti ritenete di aumentare i costi d'impresa e la pressione fiscale, perché è chiaro che gli adempimenti li fa chi paga le tasse. È una cosa che ha davvero

la forbice tra consuntivo e preventivo è enorme e soprattutto si dice che è recupero di evasione quello che invece sono errori formali cui i cittadini poi pongono rimedio regolarmente. Quindi, dobbiamo fare bene il calcolo di ciò che effettivamente si prende. Un'ultima cosa, signor Presidente:

quando ci sono maggiori entrate, quindi anche quelle derivanti dalla lotta all'evasione, si ha l'obbligo - l'ha detto poco fa la senatrice Bulgarelli - di metterli in un fondo *ex

per cui con le maggiori entrate finanziamo nuove spese. Ecco perché, altro che zero virgola! Queste sono le manovre che poi non solo irritano le Commissioni europee che sorvegliano i nostri conti (che è già una cosa importante ma non è quella decisiva), perché non riducono i fattori strutturali che abbassano la produttività del sistema Italia. Questo è il punto di fondo. E perché mi irrita? Perché è il Governo che viola deliberatamente una norma, peraltro rafforzata, come la legge di contabilità.

vituperato Senato, approva sistematicamente quella famosa deliberazione a maggioranza assoluta in cui si discute di saldo strutturale e dato che l'Italia non riesce a mantenere gli impegni sul saldo strutturale, vorrei sapere dal vice ministro Casero,

avremo conoscenze molto precise e mi auguro, anzi sono certo, che il Governo darà una risposta molto puntuale a quanto richiesto.

ho presentato una interrogazione che riguarda l'annosa vicenda di Ustica. In tale interrogazione ho richiamato, prendendola dal bollettino ufficiale della Camera, una risposta ad una interrogazione che l'allora Ministro della difesa Sergio Mattarella diede sull'argomento e naturalmente ho riportato il testo.

cosa che forse succedeva sull'Enciclopedia sovietica quando cancellavano le figure dei personaggi e dei politici caduti in disgrazia. In questo caso non c'è alcun riferimento polemico: si ricorda solo che il ministro *pro tempore* di allora, Mattarella, rispose in Parlamento sulla questione Ustica in una determinata maniera. Ora, non vorrei che passasse l'interrogazione senza il nome del Ministro e poi io dovessi collegare l'intervento svolto in Aula ricordando che il Ministro *pro tempore* che intervenne nel 2000, rispondendo all'interrogazione, era Sergio Mattarella, e fare il collegamento per far capire a coloro che leggono l'interrogazione di chi stiamo parlando. Ho trovato precedenti, sia alla Camera che al Senato, dove in interrogazioni e interpellanze, essendo presidente della Repubblica Ciampi, veniva segnalato il suo nome quando parlava, per esempio, come Presidente del Consiglio o Ministro del tesoro. Ci sono tutte le interrogazioni fatte dal Gruppo del PCI, che addirittura chiese l'*impeachment* di Francesco Cossiga quando era Capo dello Stato e quindi si rivolgeva direttamente al Capo dello Stato con parole pesantissime, chiedendone le dimissioni, e vennero accettate. Ma qui non si tratta di nulla di tutto questo. Si tratta di sapere perché, dopo una settimana, questa interrogazione

nominare il Capo dello Stato, neanche quando nelle sue precedenti funzioni, svolgeva l'incarico di Ministro, allora trarremo le nostre valutazioni. Non è però accettabile che da otto giorni questa interrogazione sia ancora all'attenzione della Presidenza del Senato per ottenere una risposta.

con questo intervento di fine seduta continuo oggi al Senato una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è, o è stata, legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne. A Nubia in provincia di Trapani, si è verificato purtroppo l'ennesimo femminicidio, una donna, Anna Manuguerra, di sessant'anni, è stata uccisa con trenta coltellate dal marito. La donna, da tutti indicata come persona umile e dedita alla famiglia, più volte aveva espresso di temere per la propria vita fino ad arrivare a chiedere la separazione, pensando che questo potesse bastare ad evitare il peggio. Salgono così a ventisette le donne che ricordiamo in questa staffetta, iniziata solo il 30 giugno. L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna. Il 46,3 per cento delle donne uccise muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata. Sono in crescita anche i casi di violenza assistita. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data, cosi come nel caso della signora Anna, che ha subito per anni le angherie fisiche e morali del marito. Si tratta sempre di una violenza cieca, di una volontà di dominio da parte di chi considera la donna non come una persona bensì come un oggetto da possedere e per questo non accetta l'abbandono. Tra due giorni, il 25 novembre, ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'intervento di oggi non vuole solo ricordare le vittime del femminicidio,

uomini e donne. Riproponiamo con convinzione il nostro appello. Un appello alla Ministra con delega per le pari opportunità e al Governo tutto: la cabina di regia che si è riunita per la prima volta l'8 di settembre monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge 119. Un appello al Paese, al Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno, non possiamo più accettare questa mattanza.

TD Group di Pisa, azienda vicina al Partito Democratico, dove trecento lavoratori hanno ricevuto una lettera in cui venivano invitati a costituire comitati per il sì al *referendum* che si terrà il 4 dicembre. L'attuale maggioranza renziana non si è limitata a precarizzare il lavoro e a rendere i lavoratori ricattabili con formule come il contratto a tutele crescenti e i *voucher*, ma adesso vuole pure che i lavoratori diventino complici nel loro progetto di smantellamento della Costituzione. Non è la prima volta che il proprietario pare che abbia proprio il chiodo fisso di voler coinvolgere i propri dipendenti affinché partecipino ad eventi a favore del Partito Democratico quando sono in corso campagne elettorali: nel maggio 2015 i suoi dipendenti dovettero assistere da un comizio del candidato del PD Antonio Mazzeo, già consigliere comunale comunale a Pisa e capolista nelle elezioni. Antonio Mazzeo venne poi eletto in Consiglio regionale e adesso è diventato responsabile del comitato regionale della Toscana per il sì. Oggi il fondatore e proprietario della TD Group si mobilita ancora una volta perché i suoi dipendenti si attivino a costituire e a far costituire uno o più comitati del sì. Naturalmente, intrecci ed importanti appalti legano TD Group alla Regione Toscana e alla politica locale e casualmente il fratello di Mazzeo ha lavorato per la TD Group e l'azienda risulta coinvolta - guarda caso - nell'inchiesta su Banca Etruria. È triste constatare la foga con cui questo imprenditore trascina i propri dipendenti in questa avventura politico-elettorale targata PD; ricorda tanto il clima aziendale descritto nei film di Paolo Villaggio, dove megadirettori invitavano i dipendenti a partecipare alle più incredibili iniziative. Lo diciamo forte e chiaro da quest'Aula, signor i lavoratori meritano rispetto! Soprattutto, i lavoratori devono essere liberi di esprimere le proprie opinioni politiche! La lettera indirizzata dall'imprenditore TD Group ai propri dipendenti risulta essere inaudita e insopportabile, lesiva del diritto fondamentale dei lavoratori alla libertà di opinione. opinione. Si tratta di un'invasione di campo nella sfera privata e personale dei lavoratori in un rapporto che non è paritario e simmetrico, come quello che si instaura tra dipendente e datore di lavoro. Il fatto che dipendenti costituiscano o meno comitati per il sì

per organizzare convegni: evidentemente avevano molto da dire! Per questo ho presentato oggi un'interrogazione ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e mi riservo di presentare un apposito esposto alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza di vigilanza affinché valutino attentamente gli eventuali illeciti. Signor Presidente, grazie al cielo non tutti lavoratori si fanno comprare per una fritturina di pesce e ci sono ancora lavoratori in grado di poter denunciare. Invitiamo quindi chiunque sia sottoposto a certi ricatti a denunciare: una forza politica che li difende